trasformato in maxiemendamento, con il quale il Governo Meloni ha dato già concreto e celere riscontro ai territori alluvionati di tre Regioni: Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Le risorse stanziate sono eccezionali e senza precedenti, pari a 4 miliardi e 500 milioni. La nomina del commissario Figliuolo, cui va tutto il nostro augurio di buon lavoro, è autorevole. Siamo sicuri che gestirà questa fase di ricostruzione successiva all'emergenza con grande competenza e spirito di servizio. Con il Governo Meloni nessuno viene lasciato indietro, imprese, famiglie e cittadini, perché tutti sono al centro di questo provvedimento. A volte in Aula si susseguono degli interventi - legittimi, per carità - recitati in politichese, con il rischio talvolta di omettere i veri contenuti del provvedimento. Da amministratore pubblico ho una *forma mentis* basata sulla concretezza, per cui preferisco in questo mio intervento in discussione generale entrare nel merito per elencare alcune misure e comprenderne la reale entità. In questo provvedimento vi sono: sospensione dei termini tributari, contributivi, previdenziali e assistenziali; sospensione dei versamenti tributari derivanti dalle cartelle di pagamento; sospensione delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti urbani che graverebbero sulle famiglie; sospensione delle rate in scadenza nell'anno in corso dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni e alle Province; sospensione anche dei procedimenti civili, penali e amministrativi; concessione della possibilità al personale appartenente all'amministrazione giudiziaria di poter svolgere il proprio lavoro in forma agile. Veniamo però adesso ai numeri: 20 milioni per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche; 10 milioni per il sostegno agli iscritti all'università, con una somma aggiuntiva di 3,5 milioni attribuita all'Università di Bologna per personale dipendente, professori e ricercatori; vicinanza totale ai lavoratori dipendenti, con un'integrazione e l'istituzione di un fondo di 620 milioni per il 2023; vicinanza assoluta ai lavoratori autonomi, anche in questo caso con un'indennità *una tantum* e uno stanziamento di 253 milioni per il 2023; sostegno alle imprese, anche con l'accesso al fondo di garanzia a titolo gratuito, senza il pagamento di alcuna commissione; 100 milioni stanziati per le attività agricole, cui si aggiungono 75 milioni di euro come fondo stanziato per l'innovazione in agricoltura; otto milioni per gli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie. è la disposizione del Ministero della cultura con cui l'incremento di un euro sul costo dei biglietto d'ingresso nei luoghi della cultura andrà ad aiutare la ricostruzione di tutto il patrimonio culturale distrutto. cinque milioni di euro per gli impianti sportivi; 10 milioni di euro a sostegno delle attività turistiche ricettive; 200 milioni di euro per incrementare il fondo per le emergenze nazionali e per coprire tutti gli interventi di somma urgenza che sono stati eseguiti miliardi di euro stanziati velocemente nella fase emergenziale, cui sono stati aggiunti 2,5 miliardi per la fase della ricostruzione, il tutto in tempo *record*, un mese dagli eventi tragici, quindi una risposta eccezionale da parte del Governo. Mi rivolgo, sempre per il tramite del Presidente, alla minoranza. Avete capito tutti questi numeri? Avete preso bene gli appunti? Avevamo abituato gli italiani alle chiacchiere; noi invece preferiamo i fatti. Il Governo Meloni non lascia indietro nessuno e continua a essere presente per aiutare le popolazioni colpite a risollevarsi e a tornare competitive. siamo abituati alla coerenza. Dopo l'analisi nel merito del provvedimento, per me doverosa nei confronti di tutti i cittadini italiani che seguono con attenzione il dibattito parlamentare, vorrei però condividere con tutti voi, per il tramite del Presidente, una riflessione più politica anche in questa fase di discussione.

Come spesso accade nella nostra Regione una parte politica, in questo caso il PD, anche in una situazione eccezionale come l'alluvione, piuttosto che fare il bene dei territori, in ogni piazza e ancor più grave in ogni sede istituzionale in cui io sono presente in qualità di vice sindaco e consigliere provinciale, ha solo fatto campagna elettorale. Non capisco, lo dico non solo da parlamentare, ma soprattutto da cittadina comune, perché se al Governo si va senza vincere le elezioni, in Aula si invoca sempre senso di responsabilità e unità nazionale e, se invece al Governo ci va chi è stato eletto democraticamente, le minoranze fanno a gara per demolire le sue azioni a scapito dei cittadini. Credete davvero che i cittadini vivano ancora nel mondo delle favole? No, fatevene una ragione. Non aspettiamo risposte rispetto a quello che abbiamo posto, perché la migliore risposta l'hanno data i cittadini il 25 settembre. Ringrazio comunque, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, chi ha creato tutte queste polemiche pretestuose. Nel mio territorio, molti esponenti del PD, soprattutto nella mia provincia, piuttosto che parlare delle attività, si sono concentrati per un mese abbondante solo sul nome del commissario e, sicuramente, su questioni elettorali future che probabilmente agitano le anime all'interno del Partito Democratico. Capisco che non è facile fare la minoranza ed è ancora più difficile per chi è sempre stato in maggioranza. Sappiate che a casa nostra il popolo è sovrano, come recita la Costituzione, e quindi dal 25 settembre le scelte competono alle forze politiche di centrodestra, che hanno ricevuto il mandato direttamente dai cittadini. Viva la democrazia! Gli attacchi continui degli ultimi tempi, in realtà, per noi sono fonte di opportunità per evidenziare, con i documenti alla mano, come la Regione Emilia-Romagna, che si è sempre descritta come la prima della classe, in sintesi non ha investito nella prevenzione. Ci sono richieste di sindaci inevase negli anni e quindi il frutto è un territorio fragile, perché nessuna politica di visione e strutturale è stata portata a compimento. Nel 2011 si erano verificati gli stessi avvenimenti. Molte sono state le richieste di pulizia dei fiumi, ma nulla è stato fatto. Cito un esempio: 23 casse di espansione necessarie per il nostro territorio, ne sono state realizzate 12 e neanche completate. Nel 2011 sono esondati gli stessi fiumi, che sono poi esondati nel 2023. Quindi ha fatto bene Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, a rientrare prima dalla missione e a recarsi nei luoghi alluvionati e benissimo hanno fatto i ministri Musumeci, Lollobrigida, Urso e Zangrillo a confrontarsi con i territori. ottimo il lavoro, di cui sono molto orgogliosa, del vice ministro Galeazzo Bignami e dell'onorevole Alice Buonguerrieri, che ho avuto l'onore di accompagnare nella provincia di Rimini, per un confronto serio e diretto con i sindaci. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che, in sinergia con i sindaci, la Protezione civile, i vigili del fuoco e le Forze dell'ordine, si sono rimboccati le maniche per dare una risposta immediata a questi territori. Concludendo, signor Presidente, l'approvazione del provvedimento nonostante le numerose polemiche degli esponenti del Partito Democratico che governa la Regione Emilia-Romagna da cinquanta anni, ma che oggi è forza politica di minoranza nel Paese e non può più orientare le scelte del Governo, va nella direzione tracciata da Giorgia Meloni. Citando le sue parole, questo Governo lavora per dare risposte concrete; a volte farà scelte impopolari, ma i cittadini hanno fiducia: ci hanno votato per fare le cose necessarie e quello continueremo a fare, per l'Italia e per tutti gli italiani.

rappresentante del Governo, la collega senatrice di maggioranza ha lanciato parecchi guanti di sfida: uno per tutti, vorrei far presente che, durante il Governo Conte,

sicuramente non io - vuole mettere in discussione il fatto che quello in carica sia un Governo eletto e faccio all'Esecutivo gli auguri di miglior governo possibile nell'interesse di tutti.

oltre a dovermi preoccupare dei miei problemi, mi sono presa l'impegno di dedicarmi anche alla soluzione dei problemi altrui ed è una grossa responsabilità che un avvocato si assume.

persone. Porto questa riflessione in Aula perché una persona che decide di impegnarsi in politica in realtà si assume l'enorme responsabilità del benessere degli degli italiani, dell'Italia e anche delle relazioni internazionali. Questa maggioranza sta certamente sollevando i rappresentanti delle opposizioni da questo senso di responsabilità,

praticamente il percorso è diventato unicamerale; il bicameralismo di fatto è scomparso e quindi noi ci ritroviamo semplicemente a votare un sì o un no. ma ve ne assumete una grande a vostro carico. Rinnovo quindi l'auspicio che riusciate a fare veramente il bene dell'Italia, anche senza accettare i consigli che possono venire dalle opposizioni. Qualcuno diceva che la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio e forse, sulla base di questa citazione, voi vi state muovendo.

che finalmente sembrava aver preso atto del fatto che abbiamo un problema dal punto di vista della cura e della gestione del territorio per il rischio idrogeologico e quindi ha parlato di quello che dovrebbe essere il primo piano di prevenzione nazionale, quando in realtà tutti noi ben sappiamo che altri Governi si sono cimentati in questo piano. Lo stesso Governo Conte, con il piano "proteggi Italia", aveva stanziato 11 miliardi in tre anni proprio per prevenire

che consente di muoversi avendo conoscenza della reale situazione sul territorio. se parliamo di un piano di prevenzione del dissesto idrogeologico, dobbiamo partire innanzitutto dal riconoscimento del fatto che stiamo vivendo un periodo di crisi, che qualcuno chiama cambiamento climatico, a qualcun altro in particolare della maggioranza, ma è sotto gli occhi di tutti ed è inconfutabile quello che sta accadendo tra siccità, alluvioni, temporali e *tornado*: è evidente che qualcosa di strano sta accadendo.

è quello dovuto all'antropizzazione del territorio. Pertanto, rispetto a un evento meteorologico come quello che è avvenuto a Milano nei giorni scorsi, che è stato veramente impressionante e devastante per la violenza con cui si è manifestato,

Un piano di prevenzione, quindi non può prescindere da una valutazione degli interventi antropici che sono stati fatti sul territorio.

poi crea dei problemi. Mi chiedo pertanto che tipo di piano di prevenzione riuscirà a fare questo Governo di destra che non appoggia l'idea di preservare la natura e di considerarla un elemento importante. a capo la presidente del Consiglio Meloni? A questo punto, per carità, cambiare idea è sintomo di intelligenza, e quindi forse questa maggioranza potrebbe ritornare sulle proprie drastiche posizioni negazioniste (la parte della maggioranza che ha manifestato quest'orientamento).

il Governo a valutare l'opportunità di», compiendo, quindi, un "giro" molto largo, e sempre compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In particolare vorrei ricordare un nostro ordine del giorno

Signor Presidente, mi consenta in premessa di dire che arriverà un tempo in cui la maggioranza smetterà di fare opposizione all'opposizione. Senatore Fina, lei non era presente quando le ho dato la parola. La inviterei a essere corretto, perché potevo anche non dargliela più, visto che non si era presentato all'inizio dei lavori. Ripeto a me stesso, perché probabilmente non sono stato chiaro, che stavo esprimendo una mia opinione. PRESIDENTE. Poteva essere dichiarato decaduto, invece sta

ripeto la mia opinione, nel merito degli interventi che ho iniziato ad ascoltare, in questo dibattito e anche nei precedenti. Io spero che, a un certo punto,

Il 31 maggio in quest'Aula si svolgeva la discussione sulla legge di conversione del decreto cosiddetto siccità. Nel mentre, i territori dell'Emilia-Romagna venivano colpiti dagli eventi calamitosi che hanno generato devastazioni, lutti e gravi danni all'economia. Oggi siamo convocati a discutere e confrontarci sulla conversione del decreto-legge che il Governo ha emanato all'indomani di quegli eventi, il decreto alluvione. E anche oggi, come il 31 maggio scorso, il Paese è alle prese con fenomeni climatici estremi, che stanno causando danni e devastazioni in varie Regioni. Anzitutto, sentiamo il dovere di esprimere ancora una volta la nostra vicinanza alle comunità della Lombardia, del Friuli e del Veneto, gravemente colpite da nubifragi e grandinate, ma anche alle comunità della Sicilia e della Puglia, alle prese con gravi incendi che mettono in pericolo centri abitati, infrastrutture, persino ospedali e che hanno già causato, purtroppo, vittime e feriti. Esprimiamo la massima vicinanza e tutto il sostegno istituzionale ai Presidenti delle Regioni, ai sindaci, ai sistemi di protezione civile e assistenza alle popolazioni, alle Forze dell'ordine, ai tanti volontari e alle tante volontarie impegnati. Un grazie al sistema di Protezione civile europeo, che non fa mancare, anche in questo caso, il suo contributo essenziale di uomini e mezzi. Vorrei sottolineare questo punto perché, per la tragedia dell'Emilia-Romagna (per dai vicini Paesi all'interno del sistema di protezione comunitario sono arrivati 120 uomini e 55 mezzi dalla Slovenia, dalla Francia, dalla Slovacchia e dal Belgio), è accaduto che si è sottolineato un esempio di solidarietà e risposta comune europea, che ha fatto il paio con la forza resiliente di un popolo, quello emiliano-romagnolo, che non possiamo definire altrimenti che esemplare. La circostanza per la quale siamo di fronte, dunque, all'ennesimo decreto per affrontare l'emergenza di eventi calamitosi, nella coincidenza di un dibattito che, incidentalmente, avviene ancora una volta con un'emergenza in corso, sottolinea ancora, laddove ve ne fosse bisogno, il segno di questi tempi e la portata epocale dei fenomeni climatici estremi dei quali siamo spettatori. un terreno di confronto politico che avrebbe dovuto e dovrebbe far registrare solidarietà e convergenze tra le forze parlamentari per soluzioni condivise, confortati da una consapevolezza diffusa sull'emergenza climatica che sta colpendo il pianeta. Leggo con qualche interesse, anche in questi ultimi giorni, interviste, da Musumeci a Zaia, che tutto sommato debbono fare i conti con la realtà, anche se con fatica e con tanti "ma" e "se". Proprio su questo terreno una parte politica, quella che oggi governa il Paese e che in Europa fa riferimento alle destre nazionaliste e conservatrici, ha scelto di assumere una posizione vagamente negazionista, che nasconde la verità degli studi scientifici e si sottrae alla responsabilità della non più rinviabile conversione ecologica. Lo stigma di questa adesione ideale, sostanzialmente negazionista, e delle conseguenti azioni di Governo è disseminato in tutti i provvedimenti che via via siamo stati chiamati a discutere in quest'Aula e nella strategia complessiva del Governo Meloni. Purtroppo non fa eccezione il provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere.

miliardi per danni a beni pubblici; oltre due miliardi per circa 70 edifici privati danneggiati; circa 900 milioni per quasi 10.000 imprese danneggiate; oltre 1 miliardo per 9.300 imprese agricole colpite. Basterebbero queste poche indicazioni e la sproporzione tra le risorse annoverate e il fabbisogno reale per comprendere la portata del tutto insufficiente del provvedimento che esaminiamo. Il fabbisogno del territorio trova la sua dimensione emergenziale anche in questo caso sui numeri: 1.105 frane disseminate in 83 Comuni, a causa di una quantità di precipitazioni pari a 4 miliardi di metri cubi di acqua caduta in circa 16.000 metri quadrati. È un provvedimento insufficiente nella dimensione delle risorse messe a disposizione dei territori, ma che denuncia anche il ritardo con il quale alcune decisioni cruciali sono state assunte nei mesi che abbiamo alle spalle. È il caso innanzitutto della nomina del commissario, ricaduta dopo lunghi silenzi e ritardi da Palazzo Chigi sul generale Figliuolo, un uomo delle istituzioni verso il quale nutriamo grande stima da sempre, a differenza della presidente Meloni e del suo Governo, che solo oggi, dopo anni di attacchi per la gestione dell'emergenza Covid, riscoprono un servitore dello Stato, capace e adatto alla sfida della ricostruzione della Romagna. una scelta dunque tardiva e contraddittoria, non solo perché in contrasto con i giudizi fino a ieri pronunciati su Figliuolo e oggi smentiti, ma anche perché assunta a prescindere, e forse persino a dispetto del territorio, cioè di quelle figure istituzionali alle quali naturalmente bisogna affidarsi nella gestione commissariale laddove il Governo fosse stato in grado di evitare partigianerie miopi, superare divisioni profonde al suo interno, emanciparsi da un certo infantilismo politico su una nomina tanto delicata. Peraltro, è una nomina a commissario che evidentemente ha il carattere della transitorietà. mancanza di risorse e di strumenti, frutto delle scelte del Governo, ma anche della bocciatura di tante nostre proposte emendative che, con spirito costruttivo, dai banchi dell'opposizione abbiamo provato ad avanzare. Maggioranza e Governo hanno rispedito al mittente questo spirito e questa disponibilità al dialogo, bocciando in modo seriale emendamenti e ordini del giorno che avrebbero dato risposte concrete: una pratica già vista e denunciata dal nostro Governo per precedenti decreti-legge, come ad esempio quello dedicato all'emergenza Ischia, gestita dall'azione del Governo, simile e medesima nelle azioni parlamentari. Abbiamo detto in Commissione che ci sarebbe bisogno per questo Paese di un codice della ricostruzione, cioè di una regola uguale per tutti che preceda gli eventi drammatici e rispetto alla quale le cittadine e i cittadini possano attenersi per sapere che cosa spetta loro. Non c'è questo codice, non c'è stato nemmeno in passato: si è incardinato nella discussione parlamentare e non si è approvato. È un limite di tutti, ma il punto è che ogni volta in questi nove mesi in cui abbiamo discusso di eventi simili - purtroppo anche in questo caso - si è registrata una disparità di diritti rispetto a quello che c'è stato in passato *(Applausi)*, anche quando, pur vituperati, c'erano altri Governi, e di questo rispondete con la vostra responsabilità davanti alle cittadine e ai cittadini a partire da quelli della Romagna. Signor Presidente, colleghe e colleghi, non si può affrontare questo tema senza rivolgere un pensiero di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni colpite in Emilia-Romagna, in Umbria, nelle Marche. Vorrei qui in particolare esprimere una profonda vicinanza alle famiglie di quanti hanno perso i propri cari negli accadimenti

quasi magiche, del Governo. Era stato chiesto nell'immediato di tenere insieme emergenza e ricostruzione, perché questa era la cosa più importante da fare. Lo avevamo imparato nella nostra terra, con il terremoto, che bisogna tenere insieme emergenza e ricostruzione. Quando si parla dell'Emilia-Romagna - lo voglio dire a chi mi ha preceduto, al primo intervento che ho ascoltato - bisogna davvero mettersi una mano sulla coscienza, provare a ricordare cosa è stata l'emergenza del terremoto e misurare la capacità straordinaria di quella gente e di quelle amministrazioni

Quando parliamo di questa alluvione, noi parliamo di 1.600 chilometri quadrati di estensione dell'alluvione in Emilia-Romagna, di sette Province colpite, di due eventi alluvionali in due settimane, di quattro miliardi di metri cubi d'acqua (in una Regione che ne consuma 1,4), di 1.500 frane in 83 Comuni. Quando si parla di questa alluvione, bisogna prima di tutto, dopo aver espresso la solidarietà doverosa e necessaria (non l'ho sentita nel primo nel primo intervento, tra l'altro di una cittadina dell'Emilia-Romagna), ringraziare quanti fin dal primo momento, dopo il silenzio terribile di quella notte,

la Romagna in fiore che portiamo nel cuore, e so quanto siamo capaci di rispondere alle difficoltà con determinazione e coraggio. Lavorando insieme, noi abbiamo il senso del "noi": noi insieme. Non stiamo a guardare e non stiamo a fare polemiche, ma mettiamo mano all'aratro e lavoriamo. Profonda conoscenza del territorio e delle proprie comunità: questo hanno rivelato gli amministratori, le sindache e i sindaci che sono corsi a lavorare. Hanno lavorato e voglio ringraziare: 1.100 vigili del fuoco, che sono stati impegnati in oltre 10.000 interventi; 350 mezzi; 506 interventi nel centro di coordinamento aereo, che ha soccorso 800 persone; volontari ovunque; 8.000 tra donne e uomini del Servizio nazionale della protezione civile; 12 colonne mobili

Noi il fango l'abbiamo spalato e spaleremo anche il fango che viene buttato sotto forma di parole sull'Emilia-Romagna. Noi non siamo tranquilli e non siamo soddisfatti. Ma non è che non siamo tranquilli e non siamo soddisfatti da questa parte dell'Aula. Non sono tranquille le persone, non è tranquilla la gente dell'Emilia-Romagna, non lo sono le imprese, non lo sono i Comuni colpiti dall'alluvione. Il decreto contiene solo un terzo delle risorse necessarie a far fronte a quanto è avvenuto. Servono risposte sui rimborsi, Servono risposte sui rimborsi, sulle proroghe delle sospensioni dei pagamenti e sui cantieri. Mancano le risorse per le imprese. Abbiamo chiesto la possibilità di dare 20.000 euro subito alle attività commerciali, come bar, negozi e piccole aziende, per dare un segnale concreto di vicinanza immediata. Ma di questo non c'è nulla.

Fatevi un giro: chi verrà in Emilia-Romagna, a parte il fatto che resterà ammirato dalla capacità dei romagnoli di rimettere in pista tutto quello che serve per le vacanze degli italiani e non solo degli italiani parlerà con le persone e capirà che non basta quello che c'è in questo decreto. Non basta. Non si sentono la vicinanza e i fatti che servono. Non sono stati prorogati la sospensione dei pagamenti di bollette, le scadenze fiscali e i mutui. Non sono stati prorogati,

anche lì non c'è ancora quanto serve. Non è arrivato nulla per ora a copertura delle centinaia di interventi che i Comuni in somma urgenza hanno dovuto fare per ripristinare almeno un minimo di normalità: riapertura delle strade, messa in sicurezza del territorio, argini. Non è stato attivato il credito d'imposta che così bene aveva funzionato nella ricostruzione post terremoto. *(Applausi)*. Il tempo scorre, sono passati già due mesi; rischiamo di arrivare all'autunno impreparati; anzi, alcune zone sono già state pesantemente e nuovamente colpite dal maltempo di questi giorni. Le imprese a oggi non sanno ancora come periziare i propri danni. L'unico sostegno alle famiglie è arrivato da quell'acconto di 3.000 euro, grazie a una sperimentazione decisa dall'amministrazione regionale con la Protezione civile per la prima volta in Italia. Funziona così: basta certificare che si è in zone alluvionate e arriva un primo bonifico che salirà a 5.000 euro. Questi aiuti stanno già arrivando alle famiglie che invece in passato hanno dovuto attendere fino a un anno. In conclusione, Presidente, mettete l'Emilia-Romagna davvero nelle condizioni di poter ripartire come merita perché è la locomotiva di questo Paese e mettete il generale Figliuolo, cui oggi finalmente volete bene, nelle condizioni di fare il proprio lavoro. Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, su un provvedimento che prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali del 1° maggio. Sinceramente sarei voluto intervenire per ben altro. Sarei voluto intervenire forse per apprezzare il lavoro fatto negli anni trascorsi, per cercare di evitare, più che fronteggiare, determinate emergenze. Ci troviamo invece a dover parlare di ristorare dei danni per ricostruire aree private, infrastrutture pubbliche, sostenere imprese e famiglie che naturalmente sono state danneggiate; addirittura siamo dovuti ricorrere alla nomina di un commissario. Chissà perché siamo dovuti ricorrere alla nomina di un commissario quando forse qualcun altro avrebbe potuto assurgere a questo ruolo.

Solo ed esclusivamente per fare un'operazione a tavolino e andare a prevedere dei vincoli. Non è però con i vincoli che si risolvono i problemi idrogeologici legati alle alluvioni. Purtroppo non è così perché oltre al danno, c'è anche la beffa di quei proprietari che si trovano dei terreni a destinazione edificabile

Perché avvengono le alluvioni? Le alluvioni avvengono per via dell'esondazione di un corso d'acqua. Perché un corso d'acqua esonda? Lo fa perché ci sono gli argini in condizioni precarie, gli alvei da pulire. Forse sono questi i problemi che ci dovremmo porre. Perché gli argini sono in condizioni precarie? Forse perché ci sono i sottoboschi che sono troppo sporchi e abbandonati. Forse perché ci sono dei tagli abusivi dei boschi, che poi naturalmente provocano le frane e vanno a riempire gli alvei dei torrenti? Forse ci dovremmo allora preoccupare di di un piano che vada a prevedere la pulizia del sottobosco e qui potremmo fare ricorso alla figura, di cui abbiamo discusso qualche giorno fa, la figura dell'agricoltore custode, dando all'agricoltore la possibilità di pulire

finisce a valle. Sarebbe opportuno pensare allora a una pulizia degli alvei. Magari sarebbe opportuno eliminare un po' di materiale inerte presente negli alvei, anche perché vengono autorizzate delle cave che, come al solito, sono sempre a monte dei torrenti: naturalmente, movimentando i materiali, chiaramente quando piove l'altro materiale scende a valle. Vi devo però porre anche un altro problema: a chi compete il controllo

la manutenzione degli alvei, le Regioni devono emettere delle ordinanze nei confronti dei Comuni. C'è probabilmente un bisticcio: ci sono troppi organi che hanno competenza. Sarebbe opportuno allora individuare un organo che ha la competenza dal controllo alla gestione, dalla polizia agli interventi che si devono andare a fare, anche perché così facendo, purtroppo, mai nessuno farà manutenzione e pulizia degli argini e dei torrenti. A proposito degli inerti, ho provato a fare due conti conti alla spicciola. Provate a immaginare un torrente largo 100 metri, con una lunghezza di un chilometro, per una profondità di 5 metri - purtroppo, con il materiale arrivato nei torrenti, i letti dei fiumi si sono alzati notevolmente - e provate a fare una moltiplicazione semplicissima: abbiamo 500.000 metri quadri di materiale che, se so solo pensassimo a rivenderlo a coloro che hanno le autorizzazioni delle cave a 5 euro per metro

dei torrenti. Per fare questo la cosa principale è che bisogna assegnare la competenza solo ed esclusivamente a un ente. Certo, il Presidente del Consiglio ha detto che nei prossimi giorni faremo un piano di prevenzione idrogeologica serio, un piano di prevenzione idrogeologica serio, nel quale sicuramente non andremo a porre quei vincoli che effettivamente non servono a risolvere il problema. In quel piano andremo però a individuare un ente unico, che abbia tutte le competenze, dal controllo alla manutenzione, dalla pulizia alla gestione; così come andremo a prevedere un piano

potremmo evitare di piangerci addosso, quando purtroppo si verificheranno certi eventi e solo così molto probabilmente riusciremo a evitare di leccarci le ferite dopo che ci siamo fatti male. mi sarei aspettato oggi una riflessione del genere e non una polemica strumentale a tutti i costi, anche perché non possiamo assolutamente accettare polemiche da chi nel passato non ha fatto niente per cercare di risolvere il problema.

ci troviamo a discutere di un'emergenza reale. Questa è la novità. Sì, perché questo Esecutivo ha uno strano concetto del presupposto costituzionale di necessità e urgenza. L'ho detto più volte e lo ribadisco ancora, perché è bene ripetere le cose, visto che non vengono comprese. Lo sappiamo bene, lo abbiamo visto con i decreti Rai, INPS, carne sintetica, ponte sullo Stretto, *rave party*. Tuttavia, anche in questo caso date prova quantomeno di imperizia. Rispondete all'emergenza con settimane di ritardo e con un testo palesemente insufficiente. Per restare nel tema del provvedimento in esame, l'Italia si sta tropicalizzando, con caldo intenso e improvvise precipitazioni che mettono in ginocchio i nostri territori e il tessuto socio-economico di intere Regioni. A questo si aggiunge il fatto che viviamo in un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico, dove la cementificazione avanza a vista d'occhio. Ve ne siete accorti, vero? Almeno di questo siete consapevoli? Spero di sì. Sono passati quasi tre mesi dalle prime inondazioni e dalle prime frane che hanno colpito l'Emilia-Romagna ed è tutto ancora al punto di partenza. Le famiglie non riescono a tornare nelle proprie abitazioni, le imprese faticano a ripartire e aspettano sostegni economici per riprendere le loro attività e gli enti locali stanno facendo uno sforzo enorme, avendo già anticipato 500 milioni di euro. In passato sbandieravate facili soluzioni, ora invece improvvisate risposte. Ma a gridarvi in faccia ci sono le famiglie e i Comuni colpiti da quella terribile alluvione. Vi sembra normale che, ad oggi, per quelle famiglie, l'unico sostegno concreto, dal punto di vista economico, per meglio intenderci, sia arrivato solo dalla Regione? Stanziate dei fondi e, anziché trovare il modo per farli arrivare a destinazione il prima possibile, ne mettete buona parte nei capitoli di bilancio dei vari Ministeri, giusto così per complicare un tantino di più il tutto. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo tentato di migliorare questo testo con le nostre proposte e alcuni nostri emendamenti sono stati accolti, chiaramente, nel corso dell'esame alla Camera in quella sede. Penso ad esempio alla possibilità di prorogare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR per i Comuni. Penso all'emendamento che consentirà ai Comuni alluvionati di non perdere le risorse loro destinate dalla legge di bilancio 2019. penso alla possibilità, per artigiani e commercianti, di stipulare contratti di locazione di durata commisurata al periodo utile alla messa in sicurezza degli immobili colpiti e, quindi, inferiore a quella prevista dalla legge. In ogni caso, onorevoli colleghi, credo che con questo decreto-legge si sia persa un'occasione davvero importante. È così nella misura in cui non siete riusciti a tenere la vostra appartenenza politica fuori da questo provvedimento. Le dichiarazioni di queste settimane di Ministri e Sottosegretari restituiscono infatti l'istantanea di una maggioranza impegnata ad auto-glorificarsi, ad auto-assolversi e mai - e dico mai - pronta a fare autocritica. *(Applausi)*. è che vi spaventino le responsabilità. Stime fondate parlano di quasi nove miliardi di euro di danni. Questa è stata la richiesta avanzata e voi ne offrite meno della metà, In questo, come in altri casi, si manifesta la vostra difficoltà nel dare le risposte. Signori del Governo e della maggioranza, quando non si hanno risposte, non è colpa della domanda e nemmeno di chi la pone. Come ci ricorda un noto aforisma, «le domande non sono mai indiscrete; le risposte lo sono, a volte», e diciamo che le vostre lo sono state in maniera eccessiva. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che il sottosegretario Bignami non si fidava delle cifre fornite dal Governatore della Regione maggiormente colpita dall'alluvione. *(Applausi)*. Sottosegretario, oltre che palesemente di parte, evidenzia scarsa conoscenza della normativa di riferimento. Mi dispiace che non sia presente il sottosegretario Bignami: avrei gradito dirgli tranquillamente in viso tutto ciò. Che dire, poi, del ministro Musumeci, che a quanto pare vedremo tra qualche istante? Probabilmente avrà pensato che, se lo fanno gli altri, può farlo anche lui e e quindi con estrema disinvoltura ha risposto ai rappresentanti degli enti locali, che gli chiedevano aiuti per fronteggiare l'emergenza, che il Governo non è un bancomat. Ma vi rendete

lo stesso Ministro che, in un'intervista due giorni fa, si è vantato di aver investito, sempre da governatore, 480 milioni contro il rischio idrogeologico in Sicilia e allo stesso tempo fa parte di un Governo che impegna 14 miliardi che impegna 14 miliardi nella costruzione di un ponte su una delle sette faglie più pericolose al mondo. *(Applausi)*. Colleghi, questo provvedimento arriva in ritardo e non risponde in maniera soddisfacente alle richieste e alle giuste aspettative di chi ha subìto danni materiali e morali elevatissimi. Noi del MoVimento 5 Stelle siamo al fianco delle popolazioni colpite e abbiamo cercato in tutti i modi di aggiustare il tiro di un decreto assai deludente, specchio di un Governo che non sa e non vuole saperne di rimboccarsi le maniche e iniziare ad affrontare i problemi reali del Paese. Siete tanto impegnati a dire di essere bravi, ma non lo avete ancora dimostrato e di certo non lo avete fatto nemmeno con questo provvedimento. *(Applausi)*.

non immediatamente diretta dei fenomeni metereologici che colpiscono ciclicamente l'Italia afferiscono a molti rapporti, anche di natura privatistica, non escludendo poi le responsabilità personali che possono generare anche disastri economici superiori ai danni materiali immediatamente contabilizzati. Inizierò questo mio intervento in discussione generale ricordando come il 10 settembre del 2017, durante l'alluvione che colpì la città di Livorno, morirono otto persone, che ricordo oggi. L'ex sindaco 5 Stelle, Filippo Nogarin, è ad oggi l'unico imputato nel processo in corso. Il 13 luglio il pubblico ministero ha chiesto quattro anni di condanna per l'ex sindaco, il pm ha commentato dicendo di aver studiato quel processo in maniera assolutamente capillare e maniacale proprio per capire. Ovviamente non commento un processo in corso, anche se vi chiedo di consentirmi di rappresentare quali gravi responsabilità possano conseguire dalla titolarità di posizioni amministrative e come, prima di questo evento eccezionale, nessuna coscienza si sia altrettanto maniacalmente dedicata a studiare quanto quel mio territorio fu malamente gestito nei decenni precedenti, tollerando il mantenimento di abitazioni costruite sui greti dei corsi d'acqua, trasformatisi in quella occasione in enormi fiumi di fango; scegliendo la tombatura di modesti fiumiciattoli che in quell'occasione sono diventati, attraverso un tappo esplosivo, una scarica di massa d'acqua che si è riversata nei seminterrati di abitazioni circostanti, uccidendo purtroppo alcuni abitanti. L'acqua o il ghiaccio che cadono dal cielo purtroppo con maggiore o minore quantità hanno un funzionamento tecnico e fisiologico uguale in ogni parte del mondo. A differire sono, purtroppo, la cultura del vivere il territorio, la scelta degli stili di vita, la qualità e la volontà degli amministratori, anche quella dei giudici, che su quei fatti devono poi magari indagare. La natura stessa di imprevedibilità è alla base del principio che libera da responsabilità chi subisca un evento del genere,

della fenomenologia delle trombe d'aria e che il fenomeno non possa più essere definito eccezionale, anche qualora si ripresenti con cadenza irregolare; si esclude quindi il caso fortuito per il soggetto che si trovasse responsabilizzato a dover risarcire dei danni.

questa volta conseguente all'alluvione che ha colpito il territorio dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche. Non parlerò quindi dell'impatto del cambiamento climatico, atteso che ieri sera già alcune trasmissioni televisive ne hanno fatto un uso discutibile anche per creare sensazionalismo televisivo, mescolando notizie e informazioni in maniera molto confusa A volte questo è anche un perfetto colpevole per individuare una causa di forza maggiore - come dicevo prima - rispetto alle gravi mancanze gestionali del territorio; mancanze cui sono poi chiamati a rispondere gli amministratori del territorio. La cultura della manutenzione e della prevenzione è un'azione di buon senso, frutto dell'agire quotidiano che nei secoli precedenti era innato nelle nostre genti, poiché metabolizzato nell'esercizio di arti e mestieri, che aveva lo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse scarne e la fatica fisica. Oggi pertanto meraviglia lo stupore per alcuni risultati di ricerche scientifiche che ci notiziano di buone prassi sulle funzioni dell'apparato radicale di certi alberi o sulla capacità ombreggiante delle piante, capaci di abbattere la temperatura, come se la nostra meravigliosa opera paesaggistica di viali, parchi storici, aree verdi delle nostre città e delle nostre campagne fosse il frutto di un mero vezzo vocato al solo gusto dell'apparenza estetica. Condivido quindi le considerazioni del senatore di Fratelli d'Italia di ristabilire una sorta di orgoglio della vanga, che è quella cultura avvezza alla fatica e al rispetto delle fatiche di generazioni precedenti e di attaccamento al territorio, che si sintetizza con la proposta che ricordava il collega prima

con l'azione quotidiana dei nostri amministratori. È tuttavia certo l'effetto prodotto dall'impatto climatico, ovvero la serie di eventi conseguenti alle estreme manifestazioni meteorologiche, dalle cui conseguenze anche in questi ultimi giorni il nostro Paese ha subìto devastazioni di opposta natura, dal fuoco all'acqua, quando non siano moti tellurici. Sono queste le principali forze naturali con cui il nostro Paese ha storicamente dovuto fare i conti, senza poter sperare in una soluzione di continuità. Oggi, pertanto, noi mettiamo a disposizione per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni tosco-romagnole e marchigiane enormi capitali pubblici, unitamente alle competenze e alla rodata esperienza di un illustre commissario per l'emergenza, che ancora una volta, con la sua nomina, acclara come la struttura militare del nostro Paese sia una delle ultime aree della pubblica amministrazione capace di garantire che, alla emanazione di ordini e provvedimenti, segua una altrettanto efficace e conseguente capacità di verifica sull'esecuzione e sull'adozione di quei comandi. Si tratta di un potere di ordinanza in deroga a disposizioni di legge, una cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori. Dotiamo quindi il commissario di un'apposita contabilità speciale a lui aperta e a lui intestata, precise e dettagliate misure per la ricostruzione privata e pubblica in deroga a norme e vincoli, affidata all'asseverazione dei professionisti, con criteri puntuali e originali anche per il trattamento di materiali destinati alle discariche. In questo senso mi trovo d'accordo anche con l'opposizione quando sostiene che sarebbe utile e forse anche necessario redigere un testo unico specifico sul complesso di norme destinate ad applicarsi in casi emergenziali, come per il caso della sospensione dei termini processuali, fiscali, una precisa indicazione delle modalità per comprovare anche la natura dei danni e la loro rapida liquidazione. Alla luce del ciclico ripetersi di eventi luttuosi e devastanti è altrettanto urgente un *corpus* normativo dell'emergenza. L'emergenza alluvionale ha inoltre meravigliato tutti i cittadini per la straordinaria risposta civica dei volontari, dai quali è stato possibile misurare la forza dell'altruismo del nostro popolo, ma anche le forme di aiuto provenienti da strutture pubbliche della pubblica amministrazione: ricordavo prima la capacità militare. Ma torno a Livorno, e al caso dell'aiuto portato in Emilia-Romagna da gruppi di agenti della Polizia municipale di Livorno, che si stanno avvicendando per dare sostegno alle popolazioni colpite dall'alluvione, collaborando con la polizia locale a presiedere i comuni dell'Unione della Romagna Faentina. Il giudizio che la Lega dà di questo provvedimento è, pertanto, assolutamente positivo. Purtroppo, avremmo avuto il piacere di non dover redigere il testo in esame, di non parlare della tragedia che ha colpito quelle terre. Altresì, ripeto che questa dovrebbe essere l'occasione per inorgoglire nuovamente i territori; per riportare anche una cultura dell'operatività e dell'operosità, cercando di allontanare quelle teorie quelle teorie che, purtroppo, a volte condizionano un corretto, pragmatico e operativo attivismo delle amministrazioni locali; per diventare preparati, pronti e dotati di strumenti immediatamente applicabili per intervenire qualora - speriamo sempre più raramente - ce ne fosse bisogno.

abbiamo oggi in discussione un decreto importante, molto atteso dalla popolazione dell'Emilia-Romagna. È un decreto cui abbiamo provato a dare un nostro contributo, ma - ahimè - anche stamattina, purtroppo, nonostante gli sforzi costruttivi, abbiamo sentito parole più di polemica che concrete.

di come aiutare al meglio le popolazioni dell'Emilia-Romagna, non di come fare il processo al Partito Democratico. *(Applausi)*. Voi non dovrete rendere conto al Partito Democratico di quello che state facendo al Governo. Dovrete rendere conto ai cittadini e ho paura che sia molto peggio. Ho paura che sia molto peggio, perché conosco i cittadini dell'Emilia-Romagna, che ho avuto l'onore di amministrare per oltre quindici anni, prima da sindaco e poi da consigliere regionale. Io vi garantisco che sarà molto peggio rendere conto a loro che a noi, perché con loro le chiacchiere hanno poco posto. posto. Prima di tutto, però, siamo qui oggi, nella solennità di quest'Aula, per rendere omaggio alle vittime, alle diciassette persone che hanno perso la vita, a tutti feriti e agli sfollati, al dolore di quelle famiglie. Nella memoria di quello che è successo c'è un grande insegnamento per tutti noi, un grande monito per i decisori politici, e non solo, a fare presto e a fare bene. L'unico modo per onorare questi sacrifici, infatti, è quello di fare presto e fare bene.

E ancora una volta permettetemi di dire, senza alcuno spirito polemico, che sarebbe giusto anche riconoscere i passi in avanti che ha fatto questo Paese con l'intuizione straordinaria di Zamberletti quando istituì il sistema della Protezione civile,

sempre il meglio di questo Paese, che sa appunto stringersi, sa essere solidale, sa essere capace di enormi sacrifici quando vede le sofferenze altrui. In questo caso, io vorrei dire un grazie personale a chi comanda la Protezione civile, il dottor Curcio, e a tutti i suoi uomini, perché li ho visti all'opera in diverse situazioni. Permettetemi una nota personale. ho visti all'opera quando ero sindaco, in occasione del terremoto del 2012, e li ho visti all'opera quando avevo la delega alla protezione civile a Palazzo Chigi, in occasione del terremoto di Amatrice. Ho visto la loro capacità straordinaria di essere vicini al dolore, alla disperazione, alla tragedia e la loro capacità, giorno dopo giorno, di restituire fiducia, senso dello Stato, fiducia nelle istituzioni, che sono il vero patrimonio che non va disperso. È per questo che noi critichiamo questo decreto-legge, signora Sottosegretaria, se posso rivolgermi a lei, tramite il Presidente. Critichiamo questo decreto perché temiamo che questa sia un'occasione persa, perché mai come in questo momento la risposta è risultata inadeguata rispetto a quello che si Lo hanno detto benissimo i miei colleghi, sottolineando il fatto che non solo c'è una sproporzione enorme tra le risorse di cui necessitiamo - i due miliardi che avete detto di avere stanziato - ma in realtà questi due miliardi non ci sono: questo è il problema vero. Per chi sa leggere i bilanci - la collega che prima è intervenuta ha detto di essere stata amministratrice, quindi dovrebbe saper leggere i bilanci - questi due miliardi non sono a disposizione; sono miliardi che erano già nel bilancio dello Stato per altre questioni e non sono a disposizione per le cose di cui abbiamo bisogno immediatamente. Abbiamo bisogno immediatamente di indennizzi alle imprese e alle famiglie; abbiamo bisogno immediatamente di restituire ai Comuni i soldi per la somma urgenza. *(Applausi)*. Non c'è nulla di tutto questo.

Presidente, c'è però una questione: non so perché, ma non riesco ad abituarmi all'idea che la politica possa migliorare imitando i difetti peggiori degli altri; la politica non è imitare i difetti degli altri. Se qualcuno ha avuto il difetto di non considerare le situazioni oggettive, non è che dovete imitarlo: siete al Governo, e governate *(Applausi).* Non è che dovete ricordare gli errori. errori. È chiaro che potrei anche dirvi che il primo piano contro il dissesto idrogeologico in questo Paese l'ha fatto un Governo a guida PD e che questo piano ha consentito e consente oggi alle aree del Bisagno e dell'Arno e ad altre di non andare più sott'acqua quando piove. Potrei dirvi che sono state stanziate diverse centinaia di milioni e diversi miliardi per questi ambiti, ma invece preferirei dire che cosa possiamo fare insieme per migliorare. Innanzitutto c'era una lezione da imparare e per questo diciamo che il decreto-legge è inadeguato e insufficiente: e insufficiente: credeteci, lo vedrete con i vostri occhi tra qualche mese, quando spero che tornerete sui luoghi dell'alluvione e vedrete le facce degli emiliano-romagnoli. Allora lo capirete.

Le risposte del Governo Monti, nonostante le grandissime difficoltà, furono molto più rapide, efficaci e capaci di dare una prospettiva di ricostruzione e di sostegno: questo è il punto che vi stiamo dicendo. Attenzione, perché aver detto che due miliardi del bilancio già stanziati - cioè due miliardi che non sono aggiuntivi miliardi che non sono aggiuntivi - non sono una risposta capace di dare sostegno, sollievo e aiuto agli emiliano-romagnoli non è una critica a Fratelli d'Italia o al

quel senso di fiducia nelle istituzioni che noi abbiamo costruito dal 2012 ad oggi. Come ha detto il presidente Mattarella (non un esponente di basso livello del PD, come sono io), l'esempio della l'esempio della ricostruzione del terremoto in Emilia-Romagna è un esempio per tutto il Paese ed è stato un esempio di efficienza e di capacità di risposta. *(Applausi)*. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, certificando il fatto che in otto anni abbiamo completato la ricostruzione di un territorio devastato. Non vi stiamo dicendo che avete sbagliato a non nominare Bonaccini presidente, ma che sbagliate a delegittimarlo come presidente. *(Applausi)*. Se è vero infatti che non possiamo delegittimare un Governo regolarmente eletto dai cittadini, come il Governo Meloni, voi non potete delegittimare il Presidente della Regione, che pure è stato direttamente e non indirettamente eletto dai cittadini. *(Applausi)*. Allora occorre rispetto per le istituzioni e per chi è stato eletto, che non rappresenta solo chi lo ha eletto, ma anche coloro che sono all'opposizione. Vorrei finire come ho iniziato. Non dovrete rendere conto a noi; dovrete rendere conto ai cittadini dell'Emilia-Romagna, perché quella gente, quelle famiglie e quelle imprese, un secondo dopo aver visto il disastro abbattersi su di sé, sul proprio sul proprio futuro e sui propri figli, si sono rimboccate le maniche e hanno detto: noi ci siamo e vogliamo sapere chi è al nostro fianco. al nostro fianco. Siccome ci hanno messo il cuore, il cervello, la volontà e la capacità, temo molto che si aspettino una altrettanto rapida, efficace, sicura e seria risposta da parte del Governo e delle istituzioni, come sanno di potere contare, questo sì, sui loro sindaci, di qualunque colore. colore. Sanno di poterci contare, mentre noi oggi vi diciamo che ancora oggi questi cittadini sanno di non poter contare sul Governo italiano e questo ci preoccupa molto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il 16 maggio sono partita la mattina presto dal mio Comune, Brisighella, in provincia di Ravenna, dove sono vice sindaco, per venire a Roma. Pioveva, ma non forte. Ero preoccupata per l'allerta meteo, considerato quanto accaduto la settimana prima, ma proprio per questo ho sperato che l'allerta, addirittura rossa, fosse dovuta a un eccesso di zelo. Purtroppo non è stato così: una tempesta perfetta si è abbattuta su parte dell'Emilia e su tutta la Romagna, la mia terra, non più raggiungibile né in auto, né in treno, tanto che sono riuscita a tornare a casa solo il giovedì mattina (il 18 maggio), un po' con il treno, un po' in auto e un po' a piedi, nel senso che, per raggiungere il mio paese, ho dovuto camminare per più di tre chilometri lungo i binari della linea ferroviaria Firenze-Faenza, purtroppo chiusa per le tante frane. Ciò che ho visto, una volta arrivata, rimarrà sempre impresso nei miei occhi. Il paesaggio non era, non è e non sarà più quello di prima: colline spaccate, sanguinanti di frane, ponti e strade che non esistono più e che non sarà più possibile ricostruire nelle stesse posizioni; e poi fango, fango, tanto fango dappertutto, fiumi esondati, case e campi allagati, intere frazioni isolate. Per giorni siamo stati senza acqua e senza energia elettrica. Una tragedia che, direttamente o indirettamente, non ha risparmiato nessuno: in molti hanno perso la casa e il lavoro di una vita e ci sono state anche delle vittime. A loro, come alle vittime del maltempo di ieri e dell'altro ieri, va il nostro cordoglio e alle famiglie va la nostra vicinanza. Come se non bastasse, a tutto ciò vanno aggiunti i danni causati dalla tromba d'aria di sabato scorso in alcuni Comuni della bassa Romagna e a Ravenna. È vero che una calamità come quella che si è verificata a maggio non poteva essere evitata, visti gli eventi eccezionali per intensità e per vastità e il fatto che si sono ripetuti nell'arco di pochi giorni. Tuttavia, se si fosse fatta la dovuta prevenzione, gli effetti sarebbero stati più limitati e ridotti; ma, si sa, la prevenzione non porta voti. Siamo tutti consapevoli - come ha ribadito il ministro Musumeci - che la tropicalizzazione è arrivata in Italia più di dieci anni fa. Sappiamo tutti che oltre la metà del territorio nazionale ricade in zona sismica e quasi la totalità è a rischio frane o dissesto idrico o idrogeologico. Eppure proprio la Regione Emilia-Romagna, il cui Presidente riveste da vari anni anche la carica di commissario contro il dissesto idrogeologico e la cui ex vice presidente aveva niente meno che la delega al patto per il clima, proprio l'Emilia-Romagna si è fatta trovare impreparata. La Regione che vuole sempre primeggiare in tutto stavolta ha primeggiato per inefficienza. È inutile riempirsi la bocca con parole come patto per il clima e tutela dell'ambiente, se poi non si è in grado di mettere in atto le azioni conseguenti, a cominciare dalle più semplici, come la pulizia dei fiumi, o se poi si rimandano indietro 55 milioni al Ministero dei trasporti, perché non si è in grado di spenderli. E non importa se quei finanziamenti non erano destinati a noi, ma all'idrovia ferrarese, resta sempre il fatto che erano finalizzati alla sicurezza idraulica e non sono sono stati spesi. Presidente, contro un terremoto non si può fare nulla, ma per limitare i danni di un'alluvione invece si può fare tanto. Nessuno però si è preso la responsabilità di quanto avvenuto, anzi. Il sindaco di Lugo, per esempio, nell'intervista a un giornale locale, ha affermato che l'alluvione è stata causata in gran parte dalla crisi climatica, sottolineando quella crisi climatica che la destra continua a negare, come a voler sottintendere che la colpa è del Governo che non fa abbastanza per contrastarla. Ho citato il sindaco di Lugo perché l'intervista è uscita pochi giorni dopo l'alluvione e ho trovato veramente di cattivo gusto scegliere quel momento per iniziare la campagna elettorale per le amministrative del 2024.

non è mai decollato), quello è proprio il Governo Meloni. Ricordo, fra l'altro, che era anche un punto del programma elettorale. Quanto alla polemica circa le parole del ministro Musumeci, che ha detto che una ricostruzione non può durare anni e anni, ma deve avere un termine, che ragionevolmente potrebbe essere di nove-dieci anni, vorrei ricordare che questa frase è stata detta in tempi non sospetti (mi sembra a febbraio) nell'ambito di un disegno di legge per l'adozione di un modello unico per le ricostruzioni, proprio per facilitarle. Quel modello che auspica il senatore Fina e che il Governo Meloni farà, a differenza dei Governi precedenti. quindi di una polemica pretestuosa e strumentale, anche perché altrimenti qualcuno dovrebbe spiegare perché la struttura commissariale per il sisma è ancora in piedi dopo undici il collega senatore Barcaiuolo, delle due l'una: o fa comodo a qualcuno mantenerla o i lavori non sono ancora finiti. Mi chiedo poi perché se la sinistra, che è stata al Governo, di riffa e di raffa, ben undici anni, era così consapevole dei rischi del cambiamento climatico e degli eventi estremi che ne sarebbero potuti conseguire, non ha portato a compimento quel piano? Perché se la sinistra, che ha sempre governato in Regione, era così consapevole dei rischi, non ha costruito tutte le casse di espansione? Perché ha costruito sistematicamente, anche nelle terre definite a pericolosità idraulica, tanto da ottenere il primato fra le Regioni per consumo di suolo nelle aree alluvionali? E perché Ravenna è la seconda provincia della Regione per consumo di suolo a rischio alluvione? E ancora, perché la Regione non ha fatto manutenzione e messo in sicurezza i corsi d'acqua, i fiumi e i torrenti, alcuni dei quali, tra l'altro, già esondati nel 2011 e nel 2019, tra cui il Savio il Sillaro? E ancora: perché nel 2017 la Regione ha varato una legge urbanistica, non ancora applicata del tutto, nonostante siano passati sei anni, che a parole dice di voler limitare il consumo di suolo, ma che di fatto consente un uso del 3 per cento? L'ettaraggio previsto per l'uso rimane praticamente lo stesso degli anni precedenti *(Applausi)*, aggravando così ancora di più il bilancio delle aree impermeabili. Insomma, perché non è stato fatto tutto il possibile per limitare e ridurre gli effetti di eventi estremi? Ipotizzo una risposta: perché la sinistra in Emilia-Romagna, per fini elettorali, si accompagna ad un certo ambientalismo, spesso integralista, che non le consente mai di avere un approccio pragmatico alle cose, ma sempre ideologico. Dopo quanto successo però, pur di nascondere la polvere sotto il tappeto e distrarre l'attenzione dalle vere responsabilità, consci di non poter incolpare solo il cambiamento climatico, hanno pensato bene di tirare in ballo anche nutrie e istrici che, come noto, hanno il vizio e la brutta abitudine di scavare le tane. Sia chiaro: l'attività di escavazione crea per forza da anni. Una volta, fra l'altro, le nutrie venivano indicate come animali nocivi: oggi questo termine non si può più usare, ma bisogna utilizzare «opportunista», quanto meno negativo. Il risultato, però, non cambia: sempre danni fanno. Sono la prima a dire che sono specie che vanno contenute, ma, se certi argini fossero stati costruiti con pietrisco, cemento armato o gabbie preconfezionate, le nutrie e gli istrici avrebbero avuto più difficoltà a scavarsi le tane.

da individuare subito il rischio di fontanazzi in caso di piena e così porvi rimedio, evitando lo straripamento. Oggi, però, i servizi di bacino sul territorio non si vedono più, si sono fatti di nebbia. Signor Presidente, i romagnoli non hanno l'anello al naso e credo che sia arrivato il momento di dare loro delle risposte serie, perché la verità è che tanti danni si potevano evitare o limitare e chi ha delle responsabilità se le deve assumere e non fare a scaricabarile, nascondendosi dietro l'eccezionalità degli eventi dovuti al cambiamento climatico e alle specie fossorie.

In due soli mesi sono quindi stati stanziati quasi cinque miliardi, praticamente la metà di quanto richiesto e sempre sperando che la cifra richiesta sia stata calcolata sui danni effettivi e non pregressi *(Applausi)*, ma questo lo appurerà il commissario.

In conclusione, credo che nella mia provincia quasi tutti i Comuni abbiano potuto constatare la solidarietà in presenza del Governo. In particolare, per il mio Comune ringrazio il vice ministro Bignami, che ci è stato molto vicino. *(Applausi)*. Voglio esprimere infine la mia gratitudine anche a tutti coloro che ci hanno aiutato: la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, le associazioni di volontariato e infine, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, i nostri ragazzi, gli angeli del fango arrivati da tutta Italia (noi li chiamiamo i *burdel de paciug*, vale a dire i ragazzi del fango).

mare*. Signor Presidente, onorevoli senatori, com'è noto, martedì pomeriggio, d'intesa con la Presidenza e con i Capigruppo, sarò in Aula per riferire sulle calamità che hanno interessato la nostra Nazione da Nord a Sud

Faremo un'analisi di ciò che è avvenuto, degli interventi coordinati dal Governo e, soprattutto, delle proposte che abbiamo il dovere di avanzare e di sottoporre, seppure nella sede più appropriata nel prosieguo dell'attività dell'Assemblea, per far fronte a una condizione che diventa sempre più insostenibile. Non ho avuto il piacere di partecipare e seguire il dibattito che si è sviluppato attorno al provvedimento in esame, ma sono certo che le tematiche sono uguali a quelle che più volte abbiamo affrontato in quest'Aula e che saremo costretti ad affrontare in futuro, se non avremo tutti il coraggio di mettere da parte i pregiudizi e di sederci attorno a un tavolo, per capire cosa realmente si può fare, senza valutare quello che non è stato fatto e avrebbe potuto essere fatto: esercizio facile, ma che rischia di compromettere l'indispensabile clima di serenità,

sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 819, di conversione,

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Signor presidente, colleghi, signor ministro Musumeci, oggi in quest'Aula esaminiamo un importante provvedimento legislativo che tocca da vicino tutti i nostri territori, che purtroppo hanno ancora delle ferite aperte. Parlo in particolare dell'Emilia-Romagna e di parte dei territori della Toscana e delle Marche. Le immagini delle onde d'acqua che hanno allagato abitazioni, aziende, strade, città, le nostre campagne, provocando purtroppo morte e distruzione, sono ancora vive nelle menti e nei cuori di tutti noi. Prima di passare alla rassegna del decreto-legge, che in realtà

dove ancora una volta hanno perso la vita due persone, e le tempeste di grandine in Veneto, che hanno provocato seri anni a famiglie, aziende e a tutto il mondo dell'agricoltura. Vorrei cogliere l'occasione per dire grazie allo straordinario mondo del volontariato, ai nostri ragazzi del fango *(Applausi)*, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e chiaramente alla nostra meravigliosa Protezione civile e a tutti i suoi volontari, che proprio nelle ore più drammatiche hanno lavorato senza sosta per salvare quante più vite possibile e aiutare tutti i cittadini di quei luoghi. Il provvedimento di oggi è uno strumento di intervento che ha anche una sua natura strutturale, in quanto azione di sistema e di programmazione che guarda quindi al futuro. Sottolineo questo aspetto perché - è vero - l'Italia è un Paese bravo a gestire le emergenze, ma tante volte purtroppo si è meno bravi il giorno dopo l'emergenza e lo stesso vale per la prevenzione. Il Governo ha dato subito però le prime risposte ai territori colpiti dall'alluvione dello scorso maggio. Cito qui solo le misure più importanti come i 30 milioni per l'attuazione dei primi interventi nelle Province romagnole, i quattro milioni per i Comuni toscani e gli altri quattro milioni destinati ai Comuni marchigiani. Grazie a questo Governo e a questa maggioranza, con questo provvedimento oggi mettiamo in campo 4,7 miliardi per risollevare le popolazioni duramente colpite dagli eventi alluvionali e franosi dello scorso maggio. Mi limito qui a citare le misure più salienti: 600 milioni per i lavoratori e la cassa integrazione, 300 milioni per i professionisti e gli artigiani, 700 milioni per sostenere la produttività delle aziende, di cui 300 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici, 100 milioni di euro per applicare il regime di aiuto per le aree a crisi industriale, 10 milioni per le imprese del settore turistico e della ristorazione. Inoltre, sono stati stanziati 200 milioni per tutto il mondo agricolo, per la nostra agricoltura, per il nostro primario, con misure come ad esempio l'integrazione del reddito mensile per i lavoratori agricoli. Si è previsto, per le società e le aziende che hanno subito danni, di sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti e inoltre l'accesso agevolato al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Abbiamo stanziato, di quei 4,7 miliardi, oltre due miliardi per la ricostruzione delle infrastrutture. Fatti dunque, non chiacchiere il bello e la concretezza di questo Governo, è il linguaggio da sempre vincente, anche nei territori, del buon governo del centrodestra. Questo provvedimento però va anche oltre e si occupa del post-emergenza. Dopo l'emergenza - dicevo - c'è una seconda fase, quella della ricostruzione. Di una nuova disciplina della ricostruzione c'era assolutamente bisogno e oggi, con questo provvedimento, si compie un passo in avanti, uniformando e quindi definendo in maniera chiara, puntuale e precisa la metodologia di intervento, la metodologia di finanziamento e poi quella, altrettanto importante, della *governance*. La *governance* è affidata a una cabina di regia che, accanto al commissario straordinario, coinvolge anche il dipartimento Casa Italia, la Protezione civile, i Presidenti delle Regioni; quindi la *governance* tiene conto dei territori e delle comunità locali, consentendo così di definire le priorità, a partire dalla riapertura delle scuole, dalla risistemazione delle strade e della viabilità, al ripristino degli argini dei fiumi e alla messa in sicurezza degli alvei. Il commissario Francesco Paolo Figliuolo, a cui va tutta la nostra riconoscenza e la nostra fiducia *(Applausi)* e che gode di una stima trasversale, è una personalità pragmatica, competente e e preparata ed è già al lavoro concreto. Sta lavorando per rivedere l'elenco dei Comuni colpiti, per redigere il piano per le opere pubbliche, il piano per i beni culturali danneggiati, per gli interventi sul dissesto idrogeologico, per le infrastrutture stradali e ambientali. C'è dunque una *road map* chiara e precisa, con una visione d'insieme che è un metodo di lavoro che noi riteniamo assolutamente efficace, efficiente e, in una parola, vincente. Questo provvedimento interviene non solo sulla ricostruzione pubblica, ma anche chiaramente su quella dei privati. Valuto quindi positivamente, in questa sede, il via libera all'emendamento sulla ricostruzione privata, grazie al quale i Comuni non dovranno farsi più carico

di tutti, condiviso certamente dai territori, a cui dobbiamo dare risposte, è evitare le lungaggini e gli intoppi che si sono verificati in passato. Non a caso infatti, grazie a questo decreto, si autorizza l'applicazione immediata dell'articolo 140 del nuovo codice dei contratti pubblici, per l'esecuzione di lavori e interventi di somma urgenza connessi alle alluvioni che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna e parte delle Regioni Marche e Toscana. L'obiettivo è correre, fare presto, fare bene e dare risposte concrete. L'obiettivo è far una volta passata l'emergenza, dopo che i riflettori mediatici si sono spenti, i territori e le comunità non si sentano abbandonati. vero che noi italiani siamo i primi al mondo nel gestire le emergenze, ma dobbiamo diventare i primi al mondo anche e soprattutto nella prevenzione e nella ricostruzione.

mentre fuori da queste porte da mesi in Italia infuriano eventi climatici estremi, in questa Aula, nei miei primi nove mesi e mezzo di lavoro con questo Governo, ho assistito con sempre più incredulità, imbarazzo e impazienza alla deliberazione di atti puramente simbolici,

registra, anche solo in Italia, un forte aumento degli eventi climatici ad alta intensità e capacità distruttiva. Le soluzioni per contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico ci sono. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo da mesi alla maggioranza un confronto sano e maturo, degno di una moderna democrazia, che riesca a porre al centro dell'attenzione i bisogni e le necessità di un Paese oggi più che mai alle prese con mille difficoltà. Non è possibile risolvere problemi nuovi con strumenti vecchi; il Governo Meloni non riesce proprio a cogliere questo concetto. Prova ne è il fatto che anche oggi ci troviamo a discutere un altro provvedimento cerotto, che non punta ad affrontare il problema alla radice, ma si limita a tamponare un'emorragia che non accenna ad arrestarsi. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, oltre a essere stato presentato con il solito rituale di totale e confusionale disorganizzazione, a cui, come già detto in altre occasioni, non mi abituerò mai, risponde con notevole ritardo alle drammatiche richieste di aiuto provenienti dalle Regioni colpite da questi eventi meteorologici estremi. Si accoda al decreto siccità, anch'esso varato con ritardo rispetto alla necessità di agire tempestivamente su una problematica stabilmente presente in Italia e per il quale ci sono voluti mesi per la nomina del commissario e per l'istituzione della cabina di regia, convocata solo una volta. Anticipa altresì il decreto-legge per la tutela dei lavoratori nell'emergenza caldo, che sarà discusso in Assemblea in autunno. Nel frattempo i famosi lavoratori che volete tanto tutelare saranno cotti a puntino. Questi sono solo alcuni esempi dell'utilizzo compulsivo e disordinato dei decreti di urgenza, i quali intervengono solo quando i problemi sono già acuti. L'utilizzo della decretazione di urgenza come mezzo per arginare i danni generati da questi eventi climatici è quindi diventato obsoleto. Questo Governo sta cercando di risolvere con uno strumento emergenziale un problema ormai diventato endemico e strutturale nel nostro Paese. In questa ottica inadeguato è anche continuare a ricorrere alla nomina di specifici commissari *ad acta*, come anche questo provvedimento fa, per la gestione di qualunque situazione emergenziale; di questo passo avremo più commissari che comuni cittadini. È un metodo inappropriato, incapace di rispondere adeguatamente agli appelli e alle richieste di tutela dei cittadini e delle imprese, che più di tutti stanno scontando sulla propria pelle le conseguenze degli eventi climatici estremi, che quotidianamente viviamo e che richiedono la messa in sicurezza del territorio e delle persone che lo abitano. Cosa manca al Governo Meloni? Manca una visione politica e metodica improntata all'adeguamento del nostro Paese e ai devastanti effetti del cambiamento climatico. Queste sfide vanno affrontate con un piano unico e organico che preveda, da un lato, il contrasto e la compensazione degli impatti causati da incendi, alluvioni e frane e, dall'altro, consenta, in un'ottica di prevenzione, di ridurre le emissioni climalteranti che contribuiscono al riscaldamento globale e sono la causa principale dello scatenarsi di questi eventi estremi. Tradotto in parole povere, il fantomatico piano Mattei, come interpretato da questo Governo, che intende sfruttare le fonti fossili del gas naturale altamente climalteranti, va messo nel cassetto per lasciare posto al potenziamento delle fonti rinnovabili. Il regolamento faro in grado di sostenere l'Italia nel percorso di mitigazione e contrasto agli eventi climatici esiste: è la normativa europea sul clima (il che risponde alle sacrosante richieste dei territori, che chiedono il rafforzamento della formazione e della riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni anche locali. Inspiegabile è il motivo per cui il Governo è sordo di fronte a questa richiesta. È infatti preoccupante delegittimare gli enti territoriali interessati e le strutture tecniche locali e non c'è nessuna ragione che possa motivare la mancanza di coraggio nell'adottare un approccio inclusivo e partecipativo dal basso, che parta dai territori. Un vero controsenso, se pensiamo alle mire autonomistiche di parte del Governo. Tale regolamento europeo prevede validi strumenti in grado di mettere a terra la tematica della decarbonizzazione e la graduale diminuzione delle emissioni climalteranti, con l'istituzione di un comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici in grado di affiancare aziende, industrie e cittadini, sostenendole concretamente nel loro lavoro di rinnovamento e transizione energetica. Questa normativa è fondamentale per incardinare un'armonizzazione di tutte le politiche pubbliche all'economia circolare, massimizzando in maniera complementare i benefici della dimensione ambientale, sociale ed economica dello sviluppo. Le risorse economiche per affrontare la mitigazione degli effetti climatici ci sono: spendiamo ogni anno oltre 22 miliardi di euro in sussidi dannosi per l'ambiente, che vanno trasformati in sussidi ambientalmente favorevoli per sostenere anche le migliaia di aziende virtuose e il cambio di rotta. Ritengo frustrante dover ripetere ancora una volta il dato che l'aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi centigradi rispetto all'era pre-industriale è causa degli eventi che stanno colpendo anche il nostro Paese e che sono sotto gli occhi di tutti. È irresponsabile che colleghe e colleghi della maggioranza ci continuino a propinare ragionamenti totalmente scollati dalla realtà, mentre fuori danni ambientali, economici e sociali stanno mettendo in ginocchio la vita di interi territori. Tutto ciò è inaccettabile nel 2023. Per tutti i motivi illustrati sopra, per tutti gli irragionevoli no del Governo a un vero cambio di rotta, annuncio il nostro no alla fiducia.

di solidarietà, di rispetto e di vicinanza ai territori colpiti dalle alluvioni e più che mai in questo caso effettivamente la decretazione d'urgenza è lo strumento che l'ordinamento prevede per consentire al legislatore un intervento immediato, rapido e quanto più efficace per affrontare quella che appunto è un'emergenza.

perché si schiaccia il ruolo del Parlamento, che è pronto a fare la sua parte, a discutere, a migliorare, a integrare i provvedimenti del Governo e non deve essere delegittimato in questo modo, perché questo significa delegittimarlo. Per entrare nel merito, signor Presidente, questo è un provvedimento che riguarda l'emergenza ambientale. In questi mesi, negli ultimi anni, abbiamo visto quanto sia facile, rovinosamente facile, che un temporale si trasformi in un nubifragio, che un nubifragio si trasformi in un ciclone e che un ciclone si trasformi in un'emergenza che comporta un'alluvione, una perdita di terreni, di aziende, di attività e di case. È stato fin troppo facile assistervi nel maggio di quest'anno e adesso abbiamo l'emergenza roghi. Cosa sta succedendo al nostro Paese? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre e le risposte non possono certamente arrivare dalla decretazione d'urgenza. Oggi, con il provvedimento al nostro esame, cerchiamo di riparare i danni, di dare un aiuto economico, di dire alle popolazioni colpite le stiamo assistendo, che cerchiamo di aiutarle nella difficile fase della ricostruzione, ma ci sono danni che non possono essere riparati, con nessuna somma al mondo. Ci sono ricordi, nelle case che sono state sommerse dal fango e distrutte, che non torneranno ad esistere neanche con il risarcimento più più generoso che possiamo immaginare. Ci sono aziende in cui sono stati persi anche gli animali e le coltivazioni, che erano il frutto di sacrifici di generazioni, che non torneranno più ad essere quelle di prima. Rinasceranno, ripartiranno, ma non saranno più quelle che erano state fatte dai nonni o addirittura dagli avi, in anni ancora lontani. Ciò significa che dobbiamo lavorare sull'emergenza climatica con una legge e con una programmazione che non dovrebbe avere una prospettiva inferiore almeno ai dieci anni, perché ci vogliono almeno dieci anni per incidere sulle politiche urbanistiche del territorio, sulle politiche emergenziali, sulle politiche ambientali, per imparare un nuovo modo attraverso il quale utilizzare il nostro territorio, il nostro suolo, le nostre risorse e lasciare i vecchi modelli di sfruttamento, che come vedete sono diventati insostenibili. Questo è ciò che mi aspetto dal Governo. Oggi esprimiamo un voto di fiducia, che non è soltanto la fiducia sul provvedimento, è una fiducia, un investimento, ma soprattutto un incoraggiamento al Governo a prendere in mano questa situazione e a volerla definitivamente affrontare. Basta con la decretazione d'urgenza! Con le decretazioni d'urgenza aiutiamo le popolazioni colpite nell'immediato, ma poi cominciamo a ragionare sul futuro. Lo dobbiamo alle future generazioni, lo dobbiamo a chi abita questa terra. È per questo motivo che mi auguro che le parole che ieri il Presidente del Consiglio ha espresso proprio sull'emergenza climatica siano seguite velocemente dai fatti.

che si trovano a scendere in campo quando le città vengono sommerse dal fango o vengono lambite dal fuoco, che devono dare aiuto e sostegno ai loro cittadini, devono fare da cuscinetto e da tramite tra le istituzioni nazionali e regionali e i loro cittadini, che vanno da loro a chiedere aiuto, sostegno sostegno e soprattutto comprensione e solidarietà. Spesso sono i sindaci a incassare la rabbia, ovvero il primo sentimento dei cittadini. Questi sindaci non vanno abbandonati, vanno aiutati e sostenuti, con risorse economiche di immediato utilizzo, perché solo così, effettivamente, i territori potranno affrontare le emergenze. Il legislatore nazionale si occupi invece di programmare

Da romagnolo, ancora prima che da politico, denuncio che il Governo delle giravolte non ha fatto abbastanza sul nostro territorio.

ben sessanta giorni. È inaccettabile che si sia fatto questo percorso, perché il territorio ha bisogno che si operi con immediatezza, non si può aspettare; questa attesa è stata estenuante perché ci sono pratiche che vanno accelerate immediatamente. D'altra parte, le risorse che arrivano da questo

persone in quest'Aula ancora sostengono che i fondi del PNRR non sono sufficienti. Tuttavia settembre è vicinissimo, siamo all'inizio di agosto, il commissario straordinario sta iniziando a operare

tipo: voi vi fidereste di Schlein e compagni? Questa è campagna elettorale fatta sulle persone che soffrono! È vergognoso comportarsi così in questa fase! *(Applausi)*. Dovete venire a vedere cosa succede sul nostro territorio prima di utilizzare queste parole!

i giovani, i ragazzi che, dopo la pandemia, con tutto quello che è successo, si sono avvicinati alla nostra Regione da tutt'Italia, sono corsi nella nostra Regione, hanno dato una mano spalando il fango,

persone che non stanno affrontando correttamente il loro percorso di vita. Loro sono arrivati per primi nel nostro territorio con le pale a spalare e ad aiutare tutti. A loro va quindi il mio ringraziamento e un grandissimo abbraccio per quello che hanno fatto in quei giorni.

con le risorse degli imprenditori dei territori. Imprenditori che stanno lavorando gratis per aiutare le loro comunità. Addirittura, imprenditori e agricoltori che hanno fatto completamente allagare i loro campi per salvare le case dei loro territori.

questo decreto era stato preannunciato più volte, con visite dei rappresentanti del Governo nei territori alluvionati, dicendo che quei territori, in particolare l'Emilia Romagna, erano una locomotiva per il Paese e non potevamo permetterci di non farla ripartire. Quindi, noi ci aspettavamo Quindi, noi ci aspettavamo tantissimo da questo provvedimento che è ovviamente urgente perché vi è l'urgenza di dare soldi ai Comuni, agli imprenditori, ai cittadini che hanno perso tutto.

l'ordinaria amministrazione, figuriamoci per la ricostruzione. Se non credete ad una forza di opposizione, almeno credete a chi avete nominato commissario per la ricostruzione, impiegandovi un tempo infinito di trenta giorni *(Applausi)*, perché eravate troppo sull'obiettivo di non far emergere il nome di Stefano Bonaccini: giammai che le istituzioni possano collaborare insieme a prescindere dalle forze politiche. Avete scelto un uomo di grande livello, che ci ha aiutato e che ha salvato il Paese della pandemia, e che ora sostiene che non ci sono le risorse adeguate. Noi abbiamo assistito, in quei giorni drammatici, delle testimonianze straordinarie: i giovani del fango, i sindaci, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, gli imprenditori, i comuni cittadini rimboccarsi le maniche e cercare di salvare il salvabile. Voglio ricordare imprenditori agricoli, che hanno preferito allagare i propri campi piuttosto che vedere danneggiati i mosaici di Ravenna, e che oggi ci chiedono: ma chi ci ridarà il nostro raccolto? Chi ci darà le risorse? Di certo non si trovano qui le risorse che servono a quegli imprenditori. invece, soffermarmi su quanto accaduto successivamente, in questi giorni. Noi abbiamo avuto delle catastrofi naturali, col Nord allagato Sud: incendi che, purtroppo, non sono una catastrofe naturale ma sono volontà dell'uomo. In questi giorni, la *premier* Meloni ha dichiarato l'importanza dei cambiamenti climatici. Noi sottolineiamo con piacere il ravvedimento della *premier* Meloni, la quale, soltanto qualche settimana fa, intervenendo in una campagna elettorale straniera, quella in Spagna, a favore di Vox, dichiarava che i cambiamenti climatici non esistono e che la transizione ecologica è una sciagura. È un bel cambiamento di e noi sottolineiamo con favore che anche la *premier* Meloni si sia accorta che ci sono i cambiamenti climatici e che quindi vanno prese delle misure concrete. Quello che ci ha sorpreso è che ha annunciato il primo grande intervento relativo al dissesto idrogeologico mai preso nel nostro Paese in tutti questi anni e che finalmente vedrà la luce grazie all'intervento di questo Governo.

- come ho detto - non risponde all'emergenza di una ricostruzione di un territorio che è stato devastato e che ancora oggi vede delle frane importanti e una mobilità che non esiste. Ancora oggi i sindaci chiedono di essere ascoltati per ripristinare almeno la possibilità di muoversi all'interno di quel territorio, cosa che è ancora impedita. Non possiamo pertanto votare a favore, ma purtroppo voteremo contro, perché avremmo voluto che fossero date delle risposte più concrete a un territorio che ne ha bisogno e a persone che lo stanno chiedendo a gran voce, a prescindere dalla appartenenza politica e dalla capacità di ascolto che voi avete dimostrato. Continuano a farlo scrivendo a noi che siamo stati eletti in quei territori, chiedendoci degli aiuti concreti, perché non ne stanno vedendo; lo dicono con rammarico, perché sono abituati a piangere poco e a operare molto, ma non sono stati dati loro gli strumenti per operare. Per questi motivi, il nostro voto è profondamente contrario e auspichiamo che al più presto porrete rimedio alla mancanza di risorse per far ripartire dei territori così importanti per la nostra economia, per la nostra bellezza, per la nostra capacità di accoglienza, e che in questo momento sono molto, molto delusi dalle risposte che voi avete dato. il decreto-legge al nostro esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri dopo i gravi eventi alluvionali dell'Emilia e della Romagna.

una risposta efficace a quegli eventi tragici anche attraverso consistenti risorse economiche destinate alla ricostruzione. ricostruzione è stata affidata ad un uomo del fare, noto per essere una persona che risolve i problemi con concretezza, efficacia e onestà, il generale Figliuolo *(Applausi)*, nominato commissario straordinario alla ricostruzione. Innanzitutto vanno rilevati la tempestività del Governo e la volontà di risolvere i problemi al di fuori di ogni polemica o speculazione politica. La nomina del commissario è avvenuta in concordia con le diverse amministrazioni, compreso il presidente della Regione Bonaccini che, come tutti i governatori, è già gravato da impegni e incombenze per gestire il suo importante territorio. Tutto l'articolato è volto a dare risposte immediate e risolutive ai danni creati dalla tragica alluvione. Oltre agli interventi consueti nei casi di calamità naturale su termini e scadenze burocratiche, si sono implementate norme specifiche per iniziare la ricostruzione. Innanzitutto è stata prevista, fino a fine agosto, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi. È stato disposto il rinvio delle udienze giudiziarie che avevano scadenze a ridosso dei giorni dei tragici eventi alluvionali. Accanto a queste, ci sono le disposizioni sul lavoro agile per il personale delle amministrazioni giudiziarie, così come sono stati sospesi i procedimenti amministrativi. Si è provveduto a dare un adeguato sostegno economico alle attività didattiche, a quelle universitarie e di formazione, per farle riprendere tempestivamente. Nel settore lavoro il decreto contiene norme per riconoscere ai lavoratori gli ammortizzatori sociali e per prevedere i rinnovi dei contratti a tempo determinato; contiene inoltre misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, le cui attività sono rimaste bloccate per diversi mesi. Sono stati rafforzati gli interventi del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che costituiscono il grosso del tessuto dei territori colpiti; così come sono previste misure di sostegno alle attività agricole alluvionate. Essendo un territorio di grandi esportatori, sono previste misure che, tramite Simest, possono sostenere con appositi contributi le imprese dell'*export*. Così come sono previste la sospensione dei termini per gli adempimenti contabili e societari e la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Non mancano gli interventi per ripristinare e consolidare le strutture sanitarie e l'intera rete dell'assistenza ospedaliera e territoriale. Essendo l'Emilia e la Romagna territori ricchi di un patrimonio culturale inestimabile, si è intervenuti per assicurarne la piena tutela; così come interventi sono stati previsti per le infrastrutture sportive e per sostenere la veloce ripresa del comparto turistico, così importante soprattutto sulla parte costiera della Regione. stata rivolta anche ai Comuni, quali enti in prima fila nella gestione del ripristino dei territori, che hanno potuto beneficiare di una serie di proroghe di incombenze. Con le norme del decreto-legge n. 88, trasfuse in questo decreto, viene affrontato il tema della ricostruzione, non solo dell'Emilia-Romagna, ma anche delle zone della Toscana e delle Marche, attraverso la figura del commissario straordinario, affiancato da una cabina per il coordinamento alla ricostruzione. Viene inoltre agevolata la ricostruzione privata, con appositi contributi che verranno gestiti dal commissario Figliuolo. A sostenere l'intero importante impianto normativo sono state stanziate consistenti risorse, appostate in un apposito fondo di ricostruzione delle zone colpite: più di due miliardi quest'anno e altri miliardi (ingenti risorse) negli anni successivi, nonostante le difficoltà di bilancio. Il lavoro del commissario Figliuolo è e sarà importante; lo vedrà impegnato in compiti molto impegnativi e per questo gli facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Voglio ringraziare anche i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, tutti i volontari e la catena della solidarietà, che, come sempre, hanno profuso un grande impegno. Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia al provvedimento e alla fiducia, voglio fare un'ultima riflessione. Io sono un alluvionato del 1994 in Piemonte so che cosa vuol dire sentirsi il fango addosso. So che cosa vuol dire sentirselo anche dopo che ti sei lavato cento volte. Sembra di averlo sottopelle. So che cosa vuol dire sentire nelle narici quella puzza del giorno dopo, che non ti abbandona anche quando non c'è più. So che cosa vuol dire il proprio territorio martoriato, distrutto, ferito: prima arriva la paura di non farcela, poi la rabbia e poi la disperazione. Mi ricordo, anche se sono passati tanti anni, che la prima cosa, dopo che hai riabbracciato i parenti e gli amici, che vuoi è che torni la normalità per poter sperare di dimenticare e di andare avanti nella tua vita. *(Applausi)*. Che cosa cerchi oltre la tua comunità che sa di non potercela fare da sola? Cerchi lo Stato,

iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Signor Presidente, onorevole colleghi e colleghe, da emiliana sono orgogliosa della risposta di questo Governo a un'emergenza così importante che ha coinvolto tre Regioni: la Regione Marche, la Regione Toscana e soprattutto l'Emilia-Romagna e in particolare la Romagna. Da emiliano romagnola sono veramente orgogliosa della mia terra, della laboriosità, del pragmatismo e della voglia di ripartenza immediata che caratterizzano gli imprenditori e i cittadini emiliano romagnoli. Qualcuno in questa Aula ha detto che sono passati ottantacinque giorni dall'alluvione e questo Governo non ha fatto niente. Ricordo che pochi giorni dopo l'alluvione, il Governo ha stanziato due miliardi,

una risposta per tutti i settori: l'agricoltura, l'allevamento, il commercio, il turismo, le piccole e medie imprese, la scuola, la sanità, i dipendenti e addirittura i lavoratori autonomi. Ringrazio le Forze dell'ordine, le Forze armate, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, il personale sanitario, le associazioni. Non voglio dimenticare nessuno. Ringrazio soprattutto i giovani del fango: quei giovani che abbiamo visto tutti tutti che si sanno far su le maniche per ripristinare il proprio territorio e le proprie attività in tutti i settori. *(Applausi)*. Vanno però messe in luce le responsabilità oggettive di chi ha amministrato per decenni quel territorio e che, all'indomani dell'evento, ha immediatamente indicato nel cambiamento climatico il capo espiatorio. Al contrario, però, il World weather attribution, un istituto formato da scienziati di tutto il mondo che verifica la correlazione sussistente tra eventi naturali e cambiamenti climatici ha sbugiardato la narrazione *mainstream*. Non si può dire con certezza che l'alluvione romagnola sia stata causata dal *climate change* e dall'uomo. Nessuno mette in discussione l'esistenza di un cambiamento climatico - si badi bene - ma il punto è determinare se e fino a quando l'uomo risulta essere responsabile all'interno di questo processo. Forse si sarebbe potuto prevedere, forse nel maggior parte dell'impatto sicuramente; se però il territorio fosse stato maggiormente presidiato e preparato, le conseguenze sarebbero potute essere meno impattanti. Dobbiamo considerare che l'alluvione è - guarda caso - avvenuta in una pianura alluvionale, dove il rischio geologico è massimo. Non lo dicono la Lega o il centrodestra. Se noi andiamo direttamente a prendere la nota dell'ISPRA del 19 maggio 2023, si illustra direttamente il territorio dell'Emilia-Romagna che è potenzialmente più allagabile rispetto ad altri. Questo ce lo dice la storia. Se noi andiamo a vedere direttamente la la rete idrica che è stata costruita dal cardinale Alberoni, che io ho ripreso all'interno dell'informativa del ministro Musumeci, sicuramente dobbiamo constatare che all'epoca avevano più lungimiranza di noi. Ci sono stati dei gravi effetti di comunicazione tra chi gestisce i fiumi e i torrenti, quindi la Regione, e gli altri gestori del sistema idrico, i consorzi di bonifica e il canale emiliano romagnolo con i conseguenti conflitti di competenza e i ritardi e le inefficienze. Sempre nella nota si legge che il 14,6 per cento del territorio regionale è considerato a pericolosità elevata e molto elevata per quanto riguarda le frane. Dobbiamo allora farci una domanda, considerando soprattutto i criteri e i fattori che ricadono sotto la responsabilità delle politiche pubbliche. È soprattutto su questi aspetti che richiamo la responsabilità dell'amministrazione regionale e locale dell'Emilia-Romagna. Attribuire il disastro al cambiamento climatico è stato il tentativo delle amministrazioni per scansare ogni responsabilità. Quest'alluvione, come quella di Ischia e come tutte le altre avvenute negli anni, dimostra purtroppo una sola cosa: negli ultimi cinquant'anni non è stato fatto nulla per la manutenzione degli argini e per la pulizia dei fiumi. Preferiamo quindi preservare la natura, l'agricoltura, gli allevamenti e, soprattutto, le persone. Dobbiamo avere una visione programmatica, costruendo adeguati argini sui fiumi, dragandoli, e pulendo gli alberi, alberi, i canali, ma anche i tombini nei paesi e nelle città, nonché i boschi. Soprattutto, oltre alla manutenzione, dobbiamo fare una seria programmazione dei lavori e questo è l'importante che dev'essere fatto. Le grandinate sono imprevedibili e il terremoto è imprevedibile, mentre l'evento alluvionale è stato un disastro annunciato. Torniamo però al decreto alluvioni, un provvedimento importante del Governo, che prevede un ventaglio di interventi in più settori, con un commissario straordinario un provvedimento che indica lo stanziamento per il funzionamento della struttura pari a cinque milioni di euro per il 2023 e il 2024 e che in totale stanzia 4,5 miliardi di euro di risposte e di fondi che devono essere utilizzati per ripristinare le attività sul territorio,

20 milioni di euro per ripristinare le attività scolastiche; 10 milioni di euro, invece, sono destinati al fondo per il turismo a supporto dei porti turistici, degli stabilimenti termali e balneari, dei parchi tematici di tutto il trasporto dei viaggiatori. Infine, all'interno del decreto ci sono norme importanti per le aziende e per i liberi professionisti, l'indennità speciale per i lavoratori autonomi, la sospensione dei termini, gli aiuti per le imprese esportatrici e la sospensione dei pagamenti delle bollette. Una richiesta importante che abbiamo fatto come Lega è che le risorse stanziate in questo decreto non siano utilizzate per altre opere sul territorio che non c'entrano nulla con l'alluvione. Per questo il commissario, entro due mesi dal suo insediamento, deve fare un'analisi puntuale degli elenchi dei danni che gli enti locali hanno fatto avere all'Emilia-Romagna e che la Regione ha girato direttamente al Governo senza controllarli. Sono contenta che sia stato individuato il commissario Figliuolo, una persona con capacità manageriali, di alto profilo, che opera con pragmatismo e imparzialità come un grande militare sa fare; una persona senza sbandamenti ideologici o politici, che ascolterà tutte le esigenze, dando risposte adeguate ai vari bisogni dei territori e di chi ha subito maggiori danni.

Come Lega, però, ritengo sia necessario ripristinare la cultura della vanga, dando sostegno agli agricoltori, che sono le vere sentinelle del territorio e sanno direttamente far fronte al dissesto idrogeologico. Infine, rivolgendomi a quanti continuano a dire che è tutta colpa del cambiamento climatico, consiglio loro direttamente la cura della zappa, anche a quegli ambientalisti che deturpano i monumenti e bloccano il traffico stradale e aereo.

Presidente, ministro Calderoli, signor Sottosegretario, il ministro Musumeci, ponendo la questione di fiducia, ha correttamente ammesso di non aver avuto il piacere di ascoltare la discussione generale. Signora Presidente, per noi era un suo dovere farlo *(Applausi)*; era necessario salvaguardare la credibilità del Governo ed era necessario per salvaguardare il ruolo del Parlamento.

ma siamo di fronte a un passaggio cruciale nel nostro Paese, con costanti problematiche, come incendi che dilagano nel Mezzogiorno, ma anche incidenti climatici anomali, che colpiscono ulteriormente aree del nostro Paese già colpite come l'Emilia-Romagna, ma anche Regioni e città importanti come la Lombardia e Milano. come la Lombardia e Milano. Dunque consideriamo questo dibattito particolarmente importante. Lo hanno detto molto bene i colleghi del Gruppo Partito Democratico: il senatore Delrio, la senatrice Zampa e il senatore Fina. Vogliamo iniziare esprimendo innanzitutto solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime *(Applausi)*, perché questo è per noi il primo rapporto necessario. Lo dico anche alla maggioranza e al Governo: è opportuno che in un prossimo provvedimento vi occupiate di istituire immediatamente un fondo per sostenere le famiglie delle vittime *(Applausi)*, cosa che ancora non è avvenuta. Riteniamo necessaria questa affinché questi eventi non lascino nell'indeterminatezza, nell'incertezza e nell'ulteriore solitudine famiglie che hanno pagato con la vita un prezzo enorme.

l'Emilia-Romagna è una terra che sa unire l'impegno sociale con iniziative utili ad uno sviluppo economico, capace sempre di rafforzare il senso di comunità. Sono terre dove è forte il senso di appartenenza. Ecco perché diciamo grazie alla Protezione civile, un volto importante, bello e straordinario di questo territorio. *(Applausi)*. Diciamo allo stesso tempo grazie ai tanti volontari, ai tanti cittadini e ai tanti amministratori che hanno saputo rappresentare e stare vicini ai propri cittadini, alle imprese e alle famiglie così pesantemente colpite. Non esisterebbe l'unità nazionale se non si legittimasse immediatamente il ruolo delle istituzioni territoriali, regionali e locali, che è così prezioso per salvaguardare l'unità nazionale e la credibilità delle istituzioni, richiamandoci immediatamente ai principi di leale collaborazione. Onorevoli colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia, avete una strana idea della democrazia. Non abbiamo mai messo in discussione la legittimità di questa maggioranza politica e dunque non mettiamo in discussione la legittimità del Governo italiano. allo stesso tempo vi chiediamo, nell'interesse del Paese, di non mettere in discussione la legittimità dei governi territoriali e regionali *(Applausi)*, che non appartengono al Partito Democratico, perché una volta eletti rappresentano tutti i cittadini di quel territorio. Insomma, avete una cultura che sembra a targhe alterne nel rispetto delle istituzioni democratiche e sembra più appartenere al passato, nel tentativo cioè di gestire il potere della ricostruzione per colpire un sistema territoriale sul piano politico *(Applausi)*. Continuo a pensare che questa sfida dimostri già nei fatti il suo fallimento e lo ha già dimostrato in passato. Ricordiamo che quei territori hanno un forte senso di appartenenza: se si tagliano le radici sulle quali si fonda la vita delle famiglie e delle imprese, quei territori reagiscono. Hanno già reagito anche durante altri tentativi di utilizzare una dicotomia e un'apertura di valori che vi hanno portato, nel 2015 nel 2020, a fare iniziative contro quella terra, per prenderla. Siete stati rispediti al mittente quando suonavate i campanelli, per cercare di dimostrare che

Siamo convinti che occorra, oggi più di ieri, ascoltare la scienza. L'Italia è destinata a subire maggiori danni rispetto ad altri Paesi. Basta leggere qualche

rispetto al 1880, nel mondo l'aumento medio della temperatura è stato di poco più di un grado centigrado, mentre in Italia siamo a 2,4 gradi centigradi in più; circa il 28 per cento del territorio italiano presenta già oggi segni di desertificazione cento dei Comuni è a rischio frane, alluvioni ed erosioni costiere. Siamo cioè in presenza di un dissesto idrogeologico che riguarda tutto il Paese. Se parliamo poi della siccità, il volume dei ghiacciai alpini si è ridotto del 50 per cento negli ultimi decenni.

dovete abituarvi ad assumervi la responsabilità che comporta essere in maggioranza e al governo del Paese, cioè affrontare le sfide. Rinunciate al costante tentativo di fare opposizione al passato e cominciate ad assumervi le responsabilità per il presente e per il futuro. Fermate prima di tutto gli apprendisti stregoni che in molti casi abitano ancora nel vostro Governo e nella vostra maggioranza: ogni giorno sentiamo dibattiti assurdi considera i cambiamenti climatici come un'invenzione della sinistra o, peggio ancora, una forma estrema dell'ambientalismo radicale. Addirittura, mettete in contrapposizione la necessità che abbiamo di un adattamento ai cambiamenti climatici del nostro Paese con una necessaria iniziativa di sviluppo economico e di crescita economica dell'intero Paese.

Di fronte all'alluvione in Emilia-Romagna, dovrebbe essere prima di tutto interesse del Governo ricercare la leale collaborazione con la Regione e gli enti territoriali, perché in gioco ci sono la competitività del nostro Paese, la ripartenza, la crescita, il lavoro e la capacità di costruire coesione sociale nell'intero Paese. C'è un pezzo di PIL che, se non viene salvaguardato, rischia di abbassare le previsioni della crescita del nostro Paese, rischia cioè di essere un problema per l'intero Paese. lo chiediamo con grande chiarezza: perché non portate in quest'Aula il più rapidamente possibile il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici? *(Applausi)*. Perché non portate in quest'Aula subito, voi che siete al governo del Paese, una legge sull'uso del suolo per passare dalla cultura del consumo alla cultura della manutenzione, della rigenerazione, del rammendo? Se volete usare Se volete usare tutta la legislatura per affrontare le emergenze, vi vogliamo dire subito che rischiate di paralizzare il Paese e di spendere il doppio delle risorse necessarie per un piano per la manutenzione, il contrasto al dissesto idrogeologico e la salvaguardia della competitività economica e sociale dell'Italia. Le questioni ambientali rappresentano un'opportunità nuova per lo sviluppo economico, non un limite.

c'è bisogno di restituire il 100 per cento dei danni alle famiglie e alle imprese, affinché lo Stato dimostri vicinanza, capacità di ripartenza e rispetto delle istituzioni. La promessa del Presidente del Consiglio dei ministri non è carta straccia, segna la credibilità delle istituzioni. Non c'è una cornice economica finanziaria sufficiente per poter dare atto che la promessa del Presidente del Consiglio diventa realtà.

perché di fronte ad una calamità l'investimento in *deficit* è la migliore risposta, perché assicura un ritorno in termini di capacità di crescita, di prodotto interno lordo, di occupazione e di lavoro. Invece, restano promesse. Per pur ribadendo la totale fiducia nei confronti del commissario, che è impegnato in un'opera di ricostruzione molto importante, non possiamo garantire la fiducia ad un Governo che disattende gli impegni del Presidente del Consiglio e che non definisce ancora una cornice normativa ed economica capace di rimettere in piedi questo territorio e di restituirgli un suo diritto: le risorse

al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Consiglio, ai Ministri e ai Vice Ministri che sono venuti sul territorio, alle Forze dell'ordine, alla Protezione civile, alle Forze armate, ai volontari, ai ragazzi del fango e a tutti e a tutti i sindaci che - ne siamo consapevoli - sono intervenuti e hanno cercato di adoperarsi in tutti i modi. Il nostro ringraziamento va davvero a tutti, di qualsiasi colore politico, anche a quelli che successivamente hanno ceduto alle polemiche.

resteranno nel cuore e nella memoria degli italiani e di quel popolo; resterà la memoria di quei campi allagati, delle case piene di fango, delle aziende e dei macchinari

continuiamo a cedere sempre e soltanto alla retorica. Lo meritano quei volti e quei vestiti sporchi di fango, perché forse quel fango è stato rimosso,

però non accettiamo e non permettiamo che il cambiamento climatico diventi la foglia di fico per nascondere le responsabilità, l'inadeguatezza e l'incapacità di chi quel territorio lo doveva curare.

neghi il cambiamento climatico, così come non lo ha negato il ministro Nello Musumeci quando ha detto, in una delle sue prime dichiarazioni, che quel piano di adeguamento al cambiamento climatico che avete lasciato nei cassetti dal 2015 e che nessuno ha preso in mano va ripreso e utilizzato. Ha parlato di piano di adeguamento al cambiamento climatico. Non risponderò neanche alle accuse pervenute dal MoVimento 5 Stelle, perché gridano ancora vendetta gli 11 miliardi mai spesi del Piano proteggi Italia, il più grande piano contro il dissesto idrogeologico, soldi mai utilizzati, e, per pietà, non ricorderò i condoni di Ischia. La verità è che qualcuno doveva pulire gli alvei, qualcuno doveva contenere la fauna selvatica, qualcuno doveva realizzare le casse di espansione e qualcuno doveva contenere l'impermeabilità del suolo.

avete ignorato addirittura voi stessi, perché negli atti della Regione, nelle vostre delibere, c'era scritto che dovevate intervenire, con quelle 23 casse di espansione che qualche collega ha citato.

filosofeggiava sulla circolarità, la linearità e le strategie attuative della neutralità. Continuava a filosofeggiare su teorie lontane dai territori, perché, purtroppo, voi avete una visione del territorio, spiace dirlo,

Mi dispiace, perché, sì, la politica non è imitare i difetti degli altri. Tra l'altro, devo dire di avere apprezzato l'intervento del collega Delrio e la moderazione con cui ci avete portato qui. Purtroppo,

non avete pulito gli alvei, non avete realizzato le casse di espansione, non avete fatto il contenimento della fauna selvatica e non avete reso permeabile il suolo. Infatti, tra i tanti *record* della Regione Emilia-Romagna, anche quello di avere il suolo più impermeabilizzato d'Italia. Ed è inutile dire che avete fatto la legge sul consumo del suolo, quando il suolo era già consumato. Questa è la verità. Arriverò poi anche

non solo pretenda di indicare quale sia la soluzione, ma addirittura di dare lezioni su come dovrebbe avvenire la ricostruzione.

Credo che anche semplicemente fare un paragone con questo Governo sia abbastanza impietoso. Non è questione che la maggioranza fa opposizione all'opposizione, perché voi siete al governo e in maggioranza in quella Regione; queste sono responsabilità che avevate voi, così come vostra responsabilità era quella di aiutare il Governo a

Credo che purtroppo sia abbastanza chiaro che in una prima fase avete collaborato e vi siete travestiti da agnelli nella speranza probabilmente che Bonaccini venisse nominato commissario. Poi, quando avete capito che Bonaccini non sarebbe stato il commissario, siete tornati quello che siete, ossia lupi, e avete iniziato a speculare sulla disgrazia. *(Applausi)*. Avete iniziato a cercare di recuperare del consenso su una disgrazia che era di tutti: questa è la verità. *(Applausi)*. A un certo punto, avete iniziato ad attaccare.

il senatore deve completare l'intervento. Senatore Lisei, la prego di rivolgersi alla Presidenza e non all'opposizione, grazie.

straordinario oggi aver stanziato per gli interventi di somma urgenza 2,5 miliardi di euro. È chiaro che questi interventi non finiranno qui, ma è altrettanto chiaro che questo Governo è intervenuto, lo ha fatto in maniera celere e continuerà a stare al fianco del popolo emiliano-romagnolo, così come ha fatto in quei giorni drammatici. Voi avete perso l'occasione di dimostrare che volevate collaborare con il Governo. Avete perso l'occasione di chiedere scusa per quanto non è stato fatto in quella Regione. Avete perso l'occasione di dimostrare almeno una volta che prima vengono gli interessi degli italiani. Per noi verranno sempre prima gli interessi degli italiani. *(Applausi)*. Siamo con il commissario Figliuolo e riguardo alle ricostruzioni basta che prendiate tutti i *tweet* di Giorgia Meloni quando difendeva il commissario Figliuolo perché noi siamo sempre con l'Esercito e con le Forze dell'ordine. *(Commenti).* Prendete un *tweet* di Giorgia Meloni, se sapete aprire un *social*, e vedrete che noi siamo sempre con l'Esercito e con le Forze dell'ordine, non a correnti alternate come fate voi. Siamo sempre con le nostre Forze dell'ordine.

nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 819, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: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

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. senatore Melchiorre).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Melchiorre.

Dichiaro chiusa la votazione.

*(v. Allegato B).* Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 61. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*. *(La seduta, sospesa

finestra") sulla mancata concessione di uno spazio per il *forum* annuale di Sbilanciamoci da parte del Comune di Cernobbio,

di svolgimento del *forum* Ambrosetti, che quest'anno si terrà a Cernobbio nei giorni dal 1° al 3 settembre 2023. Si tratta in realtà di un evento che non si tiene per la prima volta. La campagna Sbilanciamoci ha promosso il *forum* a Cernobbio anche l'anno scorso; peraltro era presente l'allora ministro delle infrastrutture Giovannini e c'erano diversi esponenti della società civile e diversi esponenti di organizzazioni sindacali. Negli anni precedenti erano state promosse altre occasioni del *forum* di Cernobbio, sempre con la presenza di Ministri e di Sottosegretari, anche in sale comunali. Peraltro, stiamo parlando di una rete, che per l'appunto si chiama Sbilanciamoci, composta da 51 organizzazioni della società civile, molto attiva e molto impegnata in tutto il territorio nazionale nella solidarietà sociale, in quella internazionale, nell'educazione, nella formazione, nella tutela dell'ambiente e nella promozione della non violenza. Tra queste 51 organizzazioni ci sono l'ARCI, il WWF, Emergency, Pax Christi, Beati i costruttori di pace: in sostanza un arcipelago molto largo di organizzazioni che da molto tempo a questa parte svolgono nel nostro Paese un lavoro molto importante e - dal mio punto di vista - molto positivo. Le chiedo per l'appunto se è a conoscenza di quello che ho appena detto; se la prefettura o la questura di Como abbiamo dato indicazioni al Comune di Cernobbio di non concedere la sala per il *forum* Sbilanciamoci per i cosiddetti motivi di ordine pubblico; cosa pensa e come pensa di poter risolvere questa situazione spiacevole che si è creata, per permettere, come negli altri anni, lo svolgimento regolare del *forum* di cui ho detto. Signor Presidente, onorevoli senatori, il prefetto di Como ha acquisito elementi informativi dal Comune, dai quali risulta che l'evento oggetto del presente atto di sindacato ispettivo parlamentare - come peraltro ricordato dall'interrogante - è programmato in concomitanza con l'annuale convegno organizzato dallo Studio Ambrosetti presso l'hotel Villa d'Este di Cernobbio, dal 1° al 3 settembre prossimi. A margine e in concomitanza con l'evento, nel corso degli anni sono state organizzate iniziative in simbolica opposizione al convegno in parola. Lo scorso anno, in particolare, ha avuto luogo l'iniziativa organizzata dall'associazione Sbilanciamoci, che aveva le caratteristiche di un contro *forum* di discussione e confronto politico, che si è svolto presso i locali dell'oratorio San Giuseppe a Cernobbio. Per quanto riguarda il *forum* Ambrosetti, in analogia con le precedenti edizioni, anche quest'anno saranno pianificati attenti i servizi di vigilanza di ordine e sicurezza pubblica, nonché misure tutorie nei confronti delle personalità che interverranno. A tale scopo presso la prefettura di Como, lo scorso 21 luglio, si è svolta una prima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del sindaco, durante la quale non sono state date indicazioni dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza in merito all'iniziativa Sbilanciamoci. Tornando però alle notizie acquisite dal Comune di Cernobbio, risulta che la comunicazione di diniego dello stesso 21 luglio, riguardante l'utilizzo della sala polifunzionale a cui lei si riferisce, luogo diverso da quello richiesto l'anno scorso, fa riferimento a motivazioni riconducibili più propriamente alle esigenze di assicurare l'ordinato svolgimento del *forum* Ambrosetti a giudizio dell'amministrazione comunale. la prefettura di Como ha evidenziato che, sempre a giudizio dell'amministrazione comunale, la sala richiesta dista 800 metri dalla sede del *forum*, si trova all'interno del plesso scolastico Don Umberto Marmori e viene usata in via prioritaria per riunioni del collegio docenti, connesse alle attività scolastiche già previste e calendarizzate a partire dal 1° settembre. La stessa prefettura ha comunicato altresì che il sindaco di Cernobbio ha comunque fatto presente di essersi reso disponibile con gli organizzatori dell'iniziativa Sbilanciamoci per individuare di comune accordo un'altra struttura per ospitare l'evento. La prefettura di Como, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto dell'autonomia dell'ente locale, continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda e a supportare iniziative del Comune volte a garantire la realizzazione di tutte le manifestazioni pubbliche richieste con modalità che assolvono alle esigenze di un ordinato svolgimento delle stesse. Confido in una prossima soluzione della vicenda.

della volontà di risolvere positivamente la questione. Mi riterrò pienamente soddisfatto quando la questione sarà risolta. Spero davvero che si risolva perché capisce bene che sarebbe un precedente onestamente inaccettabile. Stiamo parlando peraltro non di una manifestazione di piazza, ma di un convegno che si fa

uno dei peggiori attentati di stampo terroristico mafioso avvenuto in Italia, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino, membro del *pool* antimafia, e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina, il ricordo delle pagine buie del nostro passato e delle scelte coraggiose che alcuni grandi persone hanno portato avanti a costo della propria vita deve essere un faro che orienta le politiche governative di contrasto alle mafie; politiche che devono prevedere un'azione integrata che affianchi alla prevenzione e alla repressione azioni sistematiche che colpiscano con sequestri e confische i beni mafiosi per destinarli a fini sociali. Nel corso degli ultimi mesi magistratura e Forze dell'ordine hanno conseguito importanti risultati, che contribuiscono ad affermare la legalità e contrastare la mafia su tutto il territorio nazionale. È fondamentale che si prosegua in questa direzione da un lato - puntando sugli organici e rafforzando i presidi di legalità e di sicurezza e - dall'altro - sottraendo alla mafia e ai mafiosi il patrimonio immobiliare per restituirgli nuova dignità, utilizzandolo soprattutto per fini sociali. Sulle pagine dei giornali di lunedì 24 luglio si legge di una vasta operazione antimafia a Foggia e provincia, dove i Carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 80 persone tra vertici affiliati e contigui della mafia foggiana, una delle più pericolose e violente organizzazioni criminali. In questi giorni il Ministro in indirizzo ha partecipato alla sottoscrizione di un accordo istituzionale tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la Regione Siciliana, finalizzato ad implementare e migliorare la gestione dei beni stessi in ambito regionale. Secondo un *report* reso noto dal TGR Piemonte, sebbene in questa Regione i beni confiscati alle mafie continuino a crescere, quasi uno su dieci non è utilizzato. di sapere se non ritenga opportuno mettere in atto le azioni necessarie al fine di incentivare e agevolare accordi con le Regioni dell'intero territorio nazionale, affinché i vari soggetti istituzionali coinvolti lavorino congiuntamente per implementare e migliorare la gestione dei beni confiscati alla mafia in ambito regionale.

e sarà sempre una priorità del Governo. Per questa ragione siamo convinti che investire in legalità e sicurezza rappresenti una premessa fondamentale per il benessere e la crescita del Paese. A tale fine il Governo agisce simultaneamente su due fronti in particolare: per un verso, intendiamo valorizzare le elevate professionalità nelle Forze di polizia, investendo risorse, sia sul piano investigativo che su quello della prevenzione, nonché rafforzando gli organici esistenti, grazie agli specifici stanziamenti della legge di bilancio per il 2023 e alle risorse che saranno richieste dal mio Dicastero in vista della prossima manovra di bilancio. Per altro verso, grazie a una legislazione di prevenzione e contrasto delle mafie assai avanzata che ha il nostro Paese, divenuto un punto di riferimento a livello internazionale, siamo impegnati nell'azione contro le infiltrazioni criminali nel tessuto economico e sociale. In questo contesto riveste rilievo strategico la confisca dei beni acquisiti illegalmente dalla criminalità organizzata, beni che possono diventare un presidio di legalità sul territorio, concorrendo al suo sviluppo e favorendo il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

lavoro dell'attuale Governo - a oggi sono stati destinati ben 1.757 immobili, con un incremento del 79 per cento rispetto all'anno precedente, con un sensibile miglioramento anche nella gestione delle aziende confiscate che impiegano diverse migliaia di persone. Per la prima volta dalla sua istituzione l'Agenzia l'Agenzia ha recentemente avviato le procedure per la destinazione diretta agli enti del terzo settore aggiudicatari di un apposito bando nazionale di ben 242 immobili. Per migliorare ulteriormente questi risultati è essenziale il programma di potenziamento dell'organico dell'Agenzia, che porterà auspicabilmente entro l'anno - al completamento della sua dotazione di personale, oggi di 200 unità, e che il Governo con il decreto-legge n. 75, attualmente in conversione in questo ramo del Parlamento, ha ulteriormente incrementato di 100 unità. lei ricordato, senatore, qualche giorno fa sono stato alla prefettura di Palermo, dove è stato sottoscritto un accordo tra l'Agenzia nazionale e la Regione Siciliana finalizzato a valorizzare i beni confiscati presenti sul territorio regionale e per l'individuazione di possibili modalità di riuso, recupero e rigenerazione urbana, anche attraverso la collocazione di presidi delle Forze di polizia. Analogo accordo era stato sottoscritto lo scorso febbraio con la Regione Calabria, mentre ieri ho personalmente presenziato alla consegna di un immobile al Comune di Cantù per destinarlo ad attività sociali. Grazie a tali strumenti viene rafforzata la cooperazione interistituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno e l'Agenzia nazionale, anche al fine di supportare gli enti locali e valorizzare i beni confiscati per finalità istituzionali e sociali. con la Regione Siciliana, analogamente a quello che ha riguardato la Regione Calabria - si inquadra in una linea di azione volta alla promozione di analoghe intese con tutte le altre Regioni, nella consapevolezza di dover affinare gli strumenti a disposizione per agevolare la fruizione dei beni. In conclusione, voglio assicurare che ogni colpo alla criminalità organizzata ci induce ad agire con sempre più determinazione, come dimostra l'imponente operazione che pochi giorni ha inferto un durissimo colpo alla mafia foggiana, una delle più pericolose e violente organizzazioni criminali del Paese.

pericolose. Sappiamo che così non è. La DIA ha parlato di come la criminalità organizzata stia cercando di prendere le *slot machine* nel metaverso e questo ci dà il senso di dove sta andando; cosa che è stata cosa che è stata confermata alla Commissione antimafia quando siamo stati a udire i vertici della FBI e della DEA negli Stati Uniti. In tale occasione ci è stato riferito che negli Stati Uniti 2 miliardi di dollari sono stati riciclati in Bitcoin su videogiochi dei nostri ragazzi.

sono stati tutti concordi nel riconoscere all'Italia quello che lei prima diceva, signor Ministro, ovvero che l'Italia ha la migliore legislazione antimafia al mondo e ha le migliori capacità investigative al mondo. Alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine va il nostro eterno ringraziamento per questa lotta che portiamo avanti come migliori al mondo, così come ci è stato riconosciuto dalle principali agenzie investigative.

di far sbarcare una parte dei 346 migranti salvati nei giorni 15 e 16 luglio in due porti diversi: Marina di Carrara e Livorno. Tutto ciò è avvenuto a una distanza considerevole dalla zona dei soccorsi, senza che fosse fornita alcuna spiegazione su questa scelta e soprattutto sui criteri di assegnazione dei porti. Peraltro, questa decisione è arrivata il giorno successivo allo sbarco di 116 di quei migranti a Lampedusa. che si è trattato di un triplo sbarco, che ha sottoposto le persone salvate, che evidentemente già vivevano una condizione di grande fragilità, a una situazione di ulteriore fragilità, sebbene fosse necessario fornire invece assistenza medica e psicologica a molte di queste persone. Tuttavia, si potrebbe dire con una battuta che c'è stata anche una "quarta rata", perché l'interminabile ed estenuante viaggio di alcuni di questi migranti non è nemmeno finito a Livorno. Infatti, 73 minori non accompagnati, di cui 15 con meno di dieci anni, uno di un anno e uno di due, scesi a terra a Livorno, hanno dovuto riprendere il viaggio in *pullman* alla volta di Taranto. È questo un giro d'Italia triste, per noi inspiegabile, che ha i caratteri della crudeltà, una crudeltà lesiva dei più elementari diritti umani. La Regione Toscana ha espresso contrarietà rispetto alla scelta di dividere in due porti, peraltro vicini, lo sbarco dei 346 migranti della Geo Barents. L'assessora regionale alla protezione civile, Monia Monni, e l'assessora regionale per il sociale, Serena Spinelli, hanno fatto una lunga dichiarazione in merito, che riporto in parte: «Dividere in due porti di sbarco rende il viaggio (...) ancora più disumano e ci impone di predisporre il nostro sistema di protezione civile solo nel porto di Carrara, rendendo estremamente difficile garantire un'adeguata accoglienza nel porto di Livorno». L'accoglienza significa, per molti di questi migranti - pensiamo alle donne e ai minori - verificare le condizioni che li hanno portati lì, anche sotto il profilo psicologico, per poi individuare lo lo strumento migliore dell'accoglienza stessa. Anche il sindaco Salvetti si è lamentato di questo frazionamento e del fatto che ci sono stati, in sei mesi, ben sei sbarchi a Livorno, una città molto lontana dalle zone di soccorso e non necessariamente attrezzata. La Regione Toscana ha predisposto un'accoglienza su un porto, con un sistema che funziona ed è efficiente e che invece riceve delle inefficienze a causa di decisioni del Governo che non riusciamo a comprendere. D'altra parte, a Lampedusa circa 9.000 persone 9.000 persone sono sbarcate in sette giorni e nell'*hotspot* di Lampedusa ci sono più di 3.000 persone, a fronte di una capienza di 400 posti. Nel 2021 sono sbarcati 67.467 migranti e nel 2023, solo a fine giugno, ne abbiamo già 60.802, quasi quanto nell'intero 2021. Nel 2022 sono stati oltre 105.000. È evidente che, quando parliamo di accoglienza, parliamo di un sistema integrato che deve essere predisposto con dei criteri anche di economicità, efficienza, esperienza e professionalità. Questo frazionamento dei porti e poi della successiva accoglienza non si comprende, anche alla luce - lo voglio ricordare, signor Ministro - dell'allegato alla convenzione SAR del 2004 che parla di *place of safety*, di luogo sicuro, nel quale vanno garantiti i sistemi di accoglienza e anche le assistenze di tipo psicologico. psicologico. Signor Ministro, chiediamo di sapere quali sono i motivi, le ragioni e i criteri per cui quei migranti siano sbarcati in posti diversi e così lontani da quelli di prima accoglienza; quali siano le condizioni dell'*hotspot* di Lampedusa e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitarne il collasso; quali iniziative intenda altresì adottare per garantire l'accoglienza adeguata dei migranti sulle coste della Toscana e infine quali sono, se esistono, dei criteri che rivelano una sistematicità nell'attribuire porti lontani a quelle imbarcazioni.

l'impatto migratorio, con evidenti ricadute sia sulla qualità dell'accoglienza che sulla gestione dei connessi servizi di ordine e sicurezza pubblica. In piena attuazione delle vigenti disposizioni normative interne e internazionali e in sinergia con tutte le amministrazioni territoriali coinvolte, il doppio sbarco dei migranti presenti sulla Geo Barents nell'occasione è stato dettato da valutazioni tecniche relative alla sicurezza della navigazione di competenza del Comando generale delle Capitanerie di porto, nonché da esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di soccorso e accoglienza dei migranti. interroganti che queste modalità sono state ritenute legittime dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito proprio dalla Geo Barents per un altro precedente caso. Più precisamente, al fine di consentire un sollecito svolgimento delle procedure sanitarie, anche a tutela delle situazioni di vulnerabilità, le operazioni di polizia e la conseguente distribuzione dei migranti sul territorio, tenuto conto della capacità ricettiva delle strutture di accoglienza dedicate, si è stabilito di far sbarcare a Marina di Carrara i richiedenti asilo destinati ai ai centri di accoglienza straordinari siti in Toscana, dando la priorità ai minori non accompagnati, ai nuclei familiari, alle donne e infine agli uomini. La prefettura di Massa, come peraltro quella di Livorno, ha poi impartito specifiche disposizioni finalizzate a garantire lo sbarco prioritario a soggetti che richiedessero immediate cure mediche, così come individuati dai sanitari dell'ufficio di sanità marittima e della Croce rossa italiana saliti a bordo. Circa Lampedusa, le evidenzio che dopo la dichiarazione dello stato di emergenza voluto dal Governo, l'affidamento della gestione dell'*hotspot* alla Croce rossa italiana, alcuni interventi strutturali e il costante e rapido *turnover* degli ospiti della struttura, grazie a procedure accelerate di cui ora si dispone, hanno consentito di superare la situazione di assoluto degrado in cui versava tale centro prima delle iniziative di questo Governo e l'assoluta inadeguata inadeguata accoglienza riservata agli ospiti. Sono presenti oggi nell'*hotspot* 408 persone su una capienza che è stata incrementata da 440 a 680 posti. Con riferimento proprio allo stato di emergenza, non posso non evidenziare come le maggiori criticità a gestire il sistema di accoglienza, la cui capacità è stata incrementata di circa il 22 per cento sul territorio nazionale, si stiano registrando proprio nelle Regioni che, non avendo espresso l'intesa come proprio la Toscana, non sono in condizioni di avvalersi delle deroghe di protezione civile ai fini di una più tempestiva attivazione delle strutture a ciò dedicate. Di contro, proprio nelle Regioni maggiormente interessate dai flussi in ingresso come la Sicilia e la Calabria, si rivela una sostanziale tenuta del sistema di accoglienza rafforzato grazie alle misure acceleratorie introdotte per effetto dello stato di emergenza.

Ci sembra che in esse ci sia una fuga da una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Nella gestione dei flussi migratori il bilancio di questo Governo è del tutto fallimentare sia sul piano dell'efficacia operativa, sia sul piano morale e umanitario. I fallimenti sulle politiche migratorie si aggiungono a quelli sull'utilizzo dei fondi del PNRR, a quelli sulla riforma del fisco, a quelli che si manifesteranno con durezza in occasione della prossima legge finanziaria, quando assisteremo - c'è da scommetterci - all'urto fragoroso tra le risorse effettivamente disponibili e una grande quantità di promesse irrealizzabili o rovinose. In materia migratoria il vostro comportamento appare viziato - spiace doverlo dire - da malafede e superficialità. La vostra propaganda pre-elettorale è stata travolta dai fatti: anche se i TG RAI li nascondono più che possono, gli arrivi via mare sono in fortissimo aumento, il sistema dell'accoglienza è quasi al collasso, le strutture sono sovraffollate e molte sul punto di scoppiare. Il dialogo e la concertazione con i Comuni e con le Regioni, indispensabili per condurre azioni serie di accoglienza e di integrazione, è ai minimi storici. Con i Comuni si sta peraltro facendo il gioco delle tre carte anche sulla sicurezza urbana; i fondi promessi non arrivano; gli annunciati aumenti di organico delle Forze dell'ordine nemmeno. Una bugia segue l'altra. I bandi per l'accoglienza, sottofinanziati per pura demagogia, vanno deserti in misura crescente; i soggetti più affidabili del terzo settore cominciano a starne alla larga, come lei saprà. Di recente Marzio Mori della Fondazione Caritas di Firenze ha ricordato che gli enti solidaristici non sono albergatori; che le persone vanno accolte con dignità; che non si tratta solo di fornire un servizio di vitto e alloggio, ma anche di fare integrazione con iniziative opportune di inserimento sociale e lavorativo attuabili solo con fondi adeguati. poi ricordato che l'accoglienza senza integrazione non è vera accoglienza ed è un pericolo per tutti, sotto ogni punto di vista, a partire da quello della sicurezza e della coesione sociale. Tuttavia, quando si è ostaggio della propria propaganda nello specifico lo slogan ad effetto è il seguente: con noi porti chiusi e meno spese per i migranti - si fa fatica ad aprire gli occhi; invece sarebbe bene cominciare ad aprirli e anche cominciare a indicare una via concreta per superare la legge Bossi-Fini con una politica strutturale di promozione dell'immigrazione legale.

Ministro, a chiederle di cambiare strada è Zaia. Signor Ministro, se non vuole ascoltare il PD, ascolti almeno il Presidente del Veneto. Tra le cose più preoccupanti vi è poi la mancanza di programmazione, a meno di non voler chiamare programmazione le telefonate *in extremis* che i prefetti verticisticamente fanno ai sindaci per prospettare l'arrivo di lì a poche ore di un certo numero di profughi e per chiedere di trovare loro in tutta fretta una sistemazione. Questa non è programmazione: è il caos non dichiarato ed è intollerabile. In ultimo, signor Ministro, vista la situazione reale, sarebbe consigliabile evitare gli eccessi retorici: presentare come un grande successo il *memorandum* con la Tunisia è stato un azzardo molto grande da parte sua e della presidente del Quell'accordo produrrà pochissimo in termini di contenimento delle partenze ed è discutibilissimo sul piano etico, perché privo di garanzie reali sul rispetto dei diritti umani di donne, uomini e bambini che fuggono dalla fame, dalla guerra e dalle persecuzioni. Avete esaltato la recente conferenza internazionale di Roma su sviluppo e migrazioni del Mediterraneo, ma anche quell'iniziativa, al di là delle buone intenzioni, è stata solo uno *spot,* che ha fatto notizia per le assenze che ha registrato più che per le decisioni concrete (praticamente nessuna) che ha prodotto. Lo stesso può dirsi dei vari sforzi che avete fatto in sede europea, invariabilmente affondati dai Governi sovranisti di cui vi proclamate grandi amici. Signor Ministro, le chiediamo ancora una volta di prendere atto che la linea che avete fin qui seguito è sbagliata e assai dannosa. Per l'ennesima volta le chiediamo un'autocritica e un mutamento di rotta... *(Brusio)*. PRESIDENTE. Colleghi,

Signora Presidente, colleghi, sottopongo oggi pomeriggio all'attenzione dell'Assemblea un tema che è centrale, perché riguarda il personale militare a salvaguardia della difesa del nostro Paese e delle nostre istituzioni istituzioni democratiche. Ringrazio il ministro della difesa Guido Crosetto per la sua presenza oggi in Aula. Come è noto, nel Consiglio dei ministri dello scorso scorso 17 luglio 2023 è stato approvato il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega n. 119 del 2022, ha rideterminato le dotazioni organiche complessive delle nostre Forze armate (Esercito italiano, Marina militare e Si prevede in particolare un incremento del personale da 150.000 a 160.000 unità. Le nostre Forze armate sono il baluardo della nostra democrazia, il custode della nostra sicurezza e, dunque, del valore della pace e della concordia. Ricordo, fra l'altro, l'impegno profuso nelle nostre comunità e nei territori: penso, ad esempio, al ruolo svolto dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, allo straordinario contributo di professionalità, generosità e umanità fornito dai nostri militari durante la pandemia per le operazioni di soccorso, per la sicurezza dei nostri cieli e dei nostri mari e in occasione delle missioni internazionali di pace. È qualcosa di straordinario, che mi commuove e che - ne sono sicuro - è e resterà scolpito per sempre nel cuore di tutti gli italiani. Siamo orgogliosi di tutto questo. Lo scenario globale oggi è sempre più complesso e richiede nuove risposte. Siamo dunque consapevoli dell'ampliamento delle competenze e dei compiti delle Forze armate, la cui stima è riconosciuta da tutti, anche e soprattutto a livello internazionale. L'ampliamento delle competenze e dei compiti, soprattutto in materia di difesa, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, è fondamentale per proteggersi da eventuali attacchi nei confronti dei nostri siti strategici e, chiaramente, per la sicurezza della nostra Repubblica. Signor Ministro, sappiamo della sua grande attenzione rispetto a tutti questi temi. Ecco perché oggi in quest'Aula vorrei chiedere, data la rilevanza dell'intervento, di voler illustrare i principali criteri di ripartizione dei volumi organici tra le Forze armate indicare quali potrebbero essere i futuri percorsi per un reale incremento dell'efficacia e dell'operatività dello strumento militare, anche alla luce del nuovo contesto internazionale.

Poli, orientato a superare gli ormai non più sostenibili effetti della riduzione imposti dalla legge n. 244 del 2012. Dal 2012 a oggi il mondo è cambiato e, purtroppo, non è cambiato in meglio. E il modo in cui è cambiato impone di cambiare anche le Forze armate. Per questo nuovo processo di revisione dello strumento militare si è voluto mettere in campo il volume organico massimo consentito dalla delega che - lo ricordo - è pari a 10.000 unità. Solo così si può determinare il passaggio del modello professionale delle Forze armate da 150.000 al nuovo modello di 160.000, ricalibrando gli organici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e attraverso l'utilizzo di risparmi di bilancio previsti dalla stessa legge n. Nel rispetto della delega, con l'intenzione di perseguire gli obiettivi di ringiovanimento dello strumento e di alta specializzazione delle professionalità - questo diceva la delega - le 10.000 unità incrementali sono state ripartite riservandone: 5.000 ai volontari, 2.659 ai sottoufficiali, 2.341 agli ufficiali, distribuite prevalentemente tra medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri logistici dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari. In tal modo abbiamo deciso di adeguare gli organici delle Forze armate sia in funzione delle rinnovate esigenze funzionali operative sia per ripianare le posizioni organiche interforze internazionali, in modo da assicurare costantemente un livello adeguato delle cosiddette componenti operative proiettabili. All'esito dell'incremento, le dotazioni organiche complessive di ciascuna forza armata risulteranno così determinate: Esercito italiano, 93.100 unità (+3.700); Marina militare, 30.050 unità (+3.250); Aeronautica militare, 36.850 unità (+3.050). Il percorso complessivo di revisione dello strumento militare non può terminare con la accennata rivalutazione quantitativa e soprattutto qualitativa degli organici, ma dovrà essere completato dall'attuazione degli altri criteri di delega contenuti nella legge n. Tra questi, di particolare rilevanza sono, ad esempio, la riforma, la razionalizzazione organizzativa e il potenziamento del sistema sanitario militare, la creazione di una riserva ausiliare dello Stato, composta da personale militare volontario dislocato sul territorio e adeguatamente addestrato, prontamente impiegabile in caso di calamità, a sostegno delle attività di protezione civile o, in forma complementare, per le attività in campo logistico della cooperazione civile e militare. Fino a oggi, l'attuazione di richiamati criteri di delega non è stata possibile per l'assenza delle coperture finanziarie. riguardo, nella riunione del Consiglio dei ministri della scorsa settimana è stato deliberato uno specifico disegno di legge, che intende rinnovare per due anni le deleghe legislative al Governo contenute nella citata legge del 2022, che scadrebbero altrimenti ad agosto e il cui esercizio è essenziale per il completamento della revisione dello strumento militare nazionale.

forze militari devono essere attente e preparate rispetto a quello che ci aspetta. Soprattutto - come diceva lei - occorre un intervento strategico anche rispetto a medici, personale sanitario, ingegneri, informatici e tutta una serie di personale in aiuto strategico soprattutto per proteggere il nostro Paese, ma anche per intervenire nei casi - li abbiamo visti, purtroppo - di calamità nelle varie parti a livello nazionale e internazionale riguarda le missioni di pace. Credo che questo sia un compito importante e fondamentale che ancora una volta le nostre Forze armate si prepararono a fare, poiché - ribadisco quello che diceva prima - sono ancora il baluardo della nostra democrazia e i custodi della nostra sicurezza. Proprio per questo, la ringrazio.

ha deliberato un decreto legislativo di grande rilevanza per il Ministero della difesa e per il personale militare, concernente il coordinamento normativo e l'inclusione nel codice dell'ordinamento militare delle disposizioni di rango primario relative all'attuazione della libertà sindacale per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare; oltre al provvedimento citato il Ministero, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge 28 aprile 2022, n. 46, che ha normato l'esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, ha avviato (e, in molti casi, definito)

Signor Presidente, onorevoli senatori, senatrice Zedda, condivido la scelta di offrire rilevanza al decreto legislativo approvato la scorsa settimana in sede preliminare dal Consiglio dei ministri, perché esso consentirà di avere un quadro normativo chiaro, univoco e soprattutto sistematicamente collocato all'interno del codice dell'ordinamento militare. di un passo importante anche sotto il profilo simbolico, perché significa e indica l'apertura di una nuova epoca per la tutela dei diritti delle donne e degli uomini in divisa. Il provvedimento ha richiesto un importante e profondo lavoro di raccordo e coordinamento legislativo tra più fonti di rango primario che in tempi diversi hanno disciplinato, prima, la rappresentanza militare e le connesse procedure di concentrazione e, adesso, le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Lo sforzo del Dicastero relativo all'attuazione della legge n. 46 del 2022, attraverso l'adozione delle numerose disposizioni discendenti di rango primario e regolamentare, è stato considerevole. Molte di queste sono già vigenti e altre sono sulla via della definitiva conclusione e dei relativi *iter* approvativi. Oltre al decreto legislativo di cui parliamo, tra i provvedimenti di maggior rilievo approvati, direttamente strumentali al concreto avvio dell'attività delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, segnalo: il decreto che disciplina le modalità di versamento alle associazioni delle quote trattenute sulla retribuzione e il decreto legislativo n. 206 del 2022 in materia di adeguamento delle procedure di contrattazione nel comparto sicurezza e difesa, nonché di istituzione dell'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Sono invece in corso di definizione altri provvedimenti necessari al concreto avvio

previsto anch'esso dalla citata legge n. 46, relativo alla definizione della disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa anche fuori dal territorio nazionale e a bordo di unità navali. Nonostante la delega scada il 27 novembre, il provvedimento non può essere ancora tecnicamente finalizzato in quanto oggi le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non sono ancora state dichiarate rappresentative e non possono pertanto esprimere il previsto parere richiesto dalla legge. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che prevede la proroga, sino a novembre 2024, del termine per l'esercizio di tale importante delega. In estrema sintesi, l'effettiva operatività delle suddette associazioni potrà verosimilmente concretizzarsi nel corso del primo trimestre del 2024, con il citato decreto del Ministro della pubblica amministrazione, una volta realizzate le seguenti condizioni: completamento e vigenza del quadro giuridico di riferimento, ma soprattutto computo degli associati e accertamento del conseguimento delle soglie percentuali di rappresentatività previste dalla legge. Caro Ministro, è stato per me molto importante poterla interrogare su questa materia, che so essere particolarmente sentita dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare. La ringrazio, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia e di tutti i lavoratori del comparto interessato. Lei, con il Governo Meloni, sta ascoltando e dando risposte concrete

*(Az-IV-RE)*. Signor Ministro, le cronache di questi giorni ci consegnano l'immagine di un Paese profondamente ferito per eventi di maltempo davvero traumatici, infliggono un colpo credo difficilmente sostenibile a quel negazionismo climatico che pure esiste e alberga in settori della sua maggioranza. A partire dalla martoriata Emilia-Romagna, passando per la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, sono moltissimi i casi di grandinate e di trombe d'aria; situazioni nelle quali ci sono stati non solo profondi danni alle cose, ma anche vittime fra i cittadini. Per non parlare del Mezzogiorno, dove il caldo da bollino rosso ha determinato situazioni insostenibili; penso a Catania e a Palermo, città assediate e isolate, in parte perfino senza la corrente elettrica e con danni davvero incalcolabili. Io mi auguro, signor Ministro, che lei riesca a far prevalere, all'interno della sua maggioranza, la consapevolezza di uno scatto in avanti, di una presa di posizione molto ferma da parte del Governo su questo fronte. Noi la interroghiamo per conoscere quale sarà il finanziamento idoneo, tempestivo e adeguato per risarcire i danni causati dai cambiamenti climatici. Sappiamo, per esempio, che in Emilia Romagna, dove abbiamo grande fiducia nel generale Figliuolo, dei nove miliardi necessari ne sono stati stanziati solo due e mezzo. Quindi, vogliamo capire quale sarà l'intervento in quella Regione. Ricordiamo l'impegno del Governo per quanto riguarda un'unica unità di missione, Italia Sicura, per far fronte al dissesto idrogeologico. Ma vorremmo anche conoscere l'opinione del Governo per quanto riguarda il piano nazionale integrato dell'energia e del clima e il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Serve, signor Ministro, un approccio di sistema e, quindi,

In merito al tema posto dagli onorevoli interroganti, è evidente la necessità di un intervento importante da parte del Governo, e quindi dello Stato, nell'affrontare in termini di prevenzione la situazione di cambiamento climatico che stiamo vivendo. Pianificazione e controllo sono le parole chiave per evitare di rincorrere l'emergenza e continuare a rammaricarsi per gli eventi estremi e contrapposti che hanno diviso l'Italia in questi giorni. Dobbiamo affrontare questa sfida definendo procedure e meccanismi rapidi e chiari, per realizzare le centinaia di opere già programmate. Posso assicurare che il Governo è già impegnato su questo fronte per garantire un coordinamento stretto fra tutti i soggetti attuatori, nella fase sia emergenziale che in quella ordinaria. La questione principale sono non i finanziamenti, ma il meccanismo e la procedura di spesa. La lunghezza degli *iter* autorizzativi, gli intrecci di competenze e la capacità degli enti locali di gestire gare complesse e onerose sono tanti fattori che in qualche modo incidono sull'effettiva capacità di spesa, la quale deve avere una solida programmazione a monte. Per questo abbiamo fortemente sostenuto il rafforzamento tecnico delle autorità di bacino distrettuali che devono garantire che gli interventi e le risorse siano inseriti in una pianificazione generale delle misure. altresì lavorando per assicurare la piena interoperabilità delle banche dati dei sistemi di monitoraggio, che consentono un quadro conoscitivo sempre aggiornato sullo stato della situazione degli interventi e un sistema integrato avanzato di previsione degli eventi. Anche attraverso l'implementazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici miriamo, tra le altre cose, alla costruzione di un contesto organizzativo incentrato su un sistema di *governance* nazionale che possa assicurare, sulla base della condivisione delle conoscenze, una maggiore coerenza e sinergia delle azioni multilivello attraverso l'individuazione

ma dobbiamo garantire un sistema di realizzazione di interventi che garantisca il rapido impegno di tutte le risorse nazionali ed europee disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico. Faccio presente, colleghi, che ci troviamo con la programmazione del Fondo sviluppo coesione 2014-2020 con un livello di spesa bassissimo, con un intreccio delle competenze tra Stato, Regioni, Province, Comuni, enti e consorzi molto difficile, che gli interroganti conoscono bene; con situazioni legate anche a vecchi meccanismi di norma - sono da rispettare, ma sono stati cambiati recentemente - che prevedono che le assegnazioni fatte a realtà regionali, anche con l'automatico commissariamento l'incarico di commissari e di presidenti di Regione, risultano in progettazione da dieci-dodici anni, e non è ancora finita la progettazione. naturalmente a fianco della programmazione del Piano nazionale adattamento climatico e in parte del PNIEC, ancorché sia sul fronte energetico, fa parte delle fa parte delle azioni per quella programmazione nazionale che proprio gli interroganti, nella loro interrogazione, citano e che è necessario proprio a livello di organizzazione del nostro Stato.

il diniego del Governo rispetto a una proposta di Azione-Italia Viva sulla costituzione immediata - una richiesta che abbiamo avanzato all'inizio della legislatura - rispetto a un'unica unità di missione. Non solo. Il sito di «la Repubblica» evidenzia un fatto che, se confermato, sarebbe estremamente grave. Dal PNRR sarebbero escluse opere legate al dissesto idrogeologico e all'idrogeno. Non solo: ci aspettiamo da lei e dal Governo parole di chiarezza rispetto alla necessità e all'urgenza di una legge italiana sul clima. clima. Essendo questa una battaglia anche culturale, vorremmo parole di chiarezza anche con riferimento al *green deal*. Abbiamo ascoltato esponenti illustri della vostra maggioranza negare i cambiamenti climatici, l'urgenza degli interventi e criticare l'Europa. i fatti di questi giorni dimostrano, se ce ne fosse bisogno, di come siano indispensabili una legge nazionale sul clima, ma anche un cambio di approccio dal punto di vista culturale. Siamo convinti che la transizione ecologica debba essere affrontata tutelando le filiere produttive, ma occorrono interventi immediati. Occorrono un approccio sistemico e un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Noi oggi non possiamo che ringraziare la Protezione civile e il Corpo dei vigili del fuoco per il lavoro straordinario che fanno *(Applausi)*, ma da lei, Ministro, ci saremmo aspettati non l'elenco delle difficoltà, che francamente conosciamo bene - chi ha fatto l'amministratore locale le conosce bene - ma uno scatto in avanti sul PNRR e soprattutto chiarezza e interventi per risarcire le popolazioni, sostenere i sindaci e dare una risposta a quella che è un'emergenza che dura da troppi giorni.

*(M5S)*. Signor Ministro, l'interrogazione trae spunto da dati inconfutabili quanto preoccupanti. Nel 2021 le emissioni globali di CO2 provenienti da fonti fossili sono aumentate di oltre il 5 per cento, tornando quasi al livello del 2019. Nel 2021 in Italia le emissioni di gas ritenute maggiormente responsabili del cambiamento climatico ammontavano a 240 milioni di tonnellate: stiamo parlando di anidride carbonica, metano e protossido di azoto. rischiamo seriamente di mancare l'obiettivo di riduzione di emissioni al 2030 per 110 milioni di tonnellate di CO2. Le chiedo dunque che cosa state facendo o che cosa avete intenzione di fare per recuperare la rotta.

L'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima è un passaggio fondamentale per delineare la politica energetica e ambientale del nostro Paese nell'obiettivo proprio della decarbonizzazione nel medio e nel lungo termine. Il PNIEC, che sarà trasmesso prossime ore al Parlamento - risulta pubblicato nella sua integrità sul sito del Ministero e quindi è in fase di trasmissione

aggiuntivi rispetto alle azioni già previste nel PNRR, così come potenziato anche da quello che sarà il nuovo capitolo REPowerEU. L'accelerazione sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica degli edifici, l'incentivazione dell'autoconsumo energetico e la decarbonizzazione dei trasporti sono tutti ambiti chiave su cui dovranno concentrarsi le politiche pubbliche dei prossimi anni,

e avere anche forme di sostegno e di incentivazione fiscale che stimolino la transizione energetica in tutti i settori. Al tempo stesso, sarà fondamentale continuare a investire sul fronte della ricerca e dello sviluppo per offrire le migliori soluzioni tecnologiche possibili al raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione. Anche l'economia circolare dovrà fornire il suo contributo con la ricerca di soluzioni che minimizzino l'uso di materie prime, oltre che i consumi del ciclo produttivo e riducano gli scarti. Il processo di decarbonizzazione dovrà procedere di pari passo con la sicurezza energetica del Paese, che dovrà aumentare la sua resilienza e autonomia nel tempo. Tale percorso è tuttavia notevolmente complesso e non si presta a soluzioni semplici o a scelte precostituite, ma richiederà misure in grado di fornire l'utilizzo di tutte le tecnologie possibili, che tengano in considerazione i vari aspetti di sostenibilità economica e sociale, nonché di compatibilità con gli obiettivi di tutela ambientale, fermo restando che il nostro Paese ha

*(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, ma non posso dichiararmi soddisfatta. So bene che lei di certo non rientra nella categoria di quanti negano i cambiamenti climatici e ce ne ha dato prova anche in questo momento. non si può dire che stiamo facendo molto, se poi, al momento di decidere, votare e prendere decisioni con dei voti, il nostro Paese si gira dall'altra parte, come è successo con la direttiva case *green* in Europa. Quindi, pare proprio che, alla consapevolezza di dover intervenire, quando lei parla di comunità energetiche rinnovabili, di economia circolare, di ricerca e di migliori tecnologie, poi non seguano azioni politiche e voti coerenti, tanto a Bruxelles, quanto in Italia Ministro, non si può dire che bisogna investire sulle rinnovabili e poi confermare l'intenzione - come avete fatto - di fare del nostro Paese l'*hub* mediterraneo del gas. Dite che il nuovo piano recentemente inviato a Bruxelles, e quindi prossimamente pubblicato sui nostri siti istituzionali, rispetti tutti i *target* fissati, addirittura faccia anche di più, ma poi evitate di parlarci delle emissioni ETS, delle auto e delle case. Sono certa che abbiamo il dovere politico e morale di essere ambiziosi sulla tutela del clima e dell'ambiente, sia per il presente che per il futuro delle nuove generazioni, esattamente come ci ricorda la nostra Costituzione.

Signor Presidente, colleghe e colleghi,

A Milano fu una strage in cui persero la vita i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e il cittadino marocchino Moussafir Driss. Tanti sono stati i feriti, sia a Milano che a Roma. Si trattava di stragismo terroristico-mafioso e da questa Aula dobbiamo mandare un abbraccio di vicinanza ai familiari e un pensiero profondo alle vittime innocenti. strategia terroristica, che seguiva le stragi di Capaci del 23 maggio, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonino Montinaro. Vi fu poi quella di via D'Amelio, in cui persero la vita, il 19 luglio, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e la settima vittima, Rita Atria, una giovane testimone di giustizia, che si suicidò il 26 luglio

comunitaria; un tentativo di minacciare e piegare lo Stato e la democrazia, finalizzato a indebolire e allentare l'azione di contrasto al crimine organizzato e la stessa legislazione antimafia e colpire il sistema democratico. Oggi si è alzata un'unica voce rigorosa, quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un piano eversivo. Ci fu però una risposta da parte di tutte le istituzioni: Parlamento, Governo, magistratura e Forze dell'ordine. Tanti sono stati i processi che hanno assicurato alla giustizia gli autori degli attentati. Il Paese e i suoi cittadini hanno difeso la libertà ed è emersa una forte coscienza collettiva, che ha condannato in maniera forte e rigorosa la disumana violenza

alla democrazia. Dobbiamo seminare memoria, per raccogliere sempre più un impegno, che dobbiamo alla nostra Repubblica. Un pensiero, signor Presidente e colleghi, lo si deve a don Luigi Ciotti, che ha dato speranza al nostro Paese, stando sempre accanto ai familiari delle vittime e accendendo sempre un faro sull'impegno antimafia nel Paese. Eppure, in questi giorni un Ministro della Repubblica lo ha definito un signore in tonaca ignorante e superficiale e ha detto anche che,

ringrazio, senatrice Rando, anche per il filo storico e logico di un ricordo che è molto significativo in quest'Aula.

La seduta è tolta